Un grande uomo, tra l'altro anche pittore, per chi non lo sapesse. Aveva una grande capacità di analisi, un'attitudine speculativa che lo ha portato a scrivere oltre 80 libri tra saggi e testi scientifici. Non intendo commemorare Pietro Barcellona, perché non l'avrebbe voluto. Ho chiesto la parola per ricordarlo, perché l'ho conosciuto nel 1976 in un convegno sulla riforma dell'ordinamento giudiziario al Centro per la riforma dello Stato, in quella che poi diventò la sua casa. Ci incontrammo in quanto eletti al Consiglio superiore della magistratura non ancora insediato. Per me era un'emozione perché Pietro Barcellona in quel momento - io ero un giovane magistrato era l'emblema dell'uso alternativo del diritto, quello che veniva chiamato giurisprudenza alternativa, per aver raccolto gli studi che erano stati fatti in un convegno svoltosi a Catania qualche anno prima. E mi colpì molto - perché in quegli anni io insegnavo all'Università Cattolica diritto privato - la sua prima attenzione alla riforma del diritto di famiglia, di cui mi occupavo come giudice. Mi disse: «Giacomo, bisogna individuare l'ampia portata delle norme, che finalmente consentono la parità nella famiglia, la parità degli affetti». era anche professore di diritto privato, e in quella veste ha sempre privilegiato la distinzione tra regole e clausole generali, ha sempre privilegiato l'interpretazione della norma per quanto può rendere, per quanto può essere applicata, preoccupato sì della condizione di coloro che sono in situazioni di disagio,

devo riconoscere che Pietro Barcellona già in quegli anni scriveva: «Ciò che mi colpiva dell'egemonia capitalistica sulla vita quotidiana era la folle pretesa di ridurre l'uomo ad una pura dimensione economica». Si può non concordare con le sue analisi (come su alcune non concordavo), ma non si può non condividere la ricerca di un modello sociale che realizzi l'uomo in quanto persona nella società.

quando, guardandomi negli occhi, mi disse: «Non è possibile». Ma l'uomo di grande umanità era nella mia stanza, mentre era già stato eletto deputato insieme ad Aldo Rizzo, in occasione di un incidente che aveva coinvolto una serie di magistrati.

scrisse: «(...) nell'idea di comunismo che avevo perseguito si manifestava un delirio di onnipotenza in cui una sorta di esplosione megalomanica tendeva ad impedire l'emersione di ogni punto di vista diverso». Era questo Pietro Barcellona: l'onestà intellettuale. Concludo, signor Presidente. Tutta la sua vita, quella che da ultimo viene chiamata la conversione al cattolicesimo di Pietro Barcellona, non è altro che un percorso, che malamente ho cercato di ripercorrere, di ripercorrere, di ricerca filosofica, che lo ha caratterizzato per tutta la vita e che può essere condensato in una delle ultime cose che ha scritto: (...) che la via della salvezza e la fuoriuscita dal pensiero unico dell'economia dominante possono realizzarsi soltanto restituendo all'uomo la sua vocazione divina». *Vale,* Pietro. *(Applausi)*.

Signor Presidente, voglio ricordare qui, oggi, Pietro Barcellona, andando oltre la definizione che ne danno le note biografiche: lo ha fatto già Giacomo Caliendo, e lo ringrazio. Pietro fu, certo, docente universitario, componente del CSM e parlamentare e per molti - anche per molti di noi Io l'ho incontrato a diciotto anni: facoltà di giurisprudenza, Catania, primo anno, corso di diritto privato. Appartengo a quella generazione di ragazzi e ragazze degli anni Settanta che avevano scelto di essere giuristi che furono educati da Pietro Barcellona ad esserlo per le strade impervie del non arrendersi alla dommatica e alla manualistica tradizionale, ma da lì partire - studiandola prima, però, profondamente per capire come il diritto potesse dare altre risposte che non quelle già date e sedimentate, come potesse continuare a conservare la propria potenza, attraverso l'interpretazione, nell'essere utile al cambiamento alla capacità di riequilibrare i rapporti economici e sociali e i rapporti di forza tra individui e gruppi, e per capire dunque come potesse essere utile per lo stesso cambiamento del Paese l'uso alternativo del diritto a cui Giacomo Caliendo ha fatto riferimento. Questa teoria lo vide protagonista e, con tutti i limiti che ha svelato, contribuì a cambiare la fisionomia e il ruolo dei giuristi italiani nella vita del Paese. Già in questo Pietro Barcellona svelò il suo non essere dommatico: in questo mai accontentarsi e nell'educare a mai accontentarsi di ciò che è dato, di ciò che è facile, troppo facile, di ciò che sembra non discutibile, perché complessa è la realtà e mutevoli i suoi rapporti. E per Pietro e per noi diventò mai esausta la ricerca di risposta. Questo tratto lo accompagnò e lo definì, e come giurista e come politico, ma potrei dire anche nelle altre forme nelle quali esercitò la sua opera di intellettuale. Qualunque fosse la questione di cui si ragionava, ciò che colpiva in lui e a cui educava era il partire dall'averla studiata assai profondamente, per poi riuscire a ripartire, cercando la verità, la risposta - non voglio usare parole improprie - con un punto di vista che niente doveva a tutto ciò che era già stato detto. C'era in questo una sorta di innocenza, un'assenza di stigma, un'assenza di crisma, che spiazzava, disorientava, irritava. Era la sua forza e la sua debolezza ed era anche la conferma che, qualunque fosse stato il campo della sua ricerca (il diritto, la filosofia, l'antropologia o la teologia), Pietro Barcellona si confermava sempre come un grande intellettuale, e certo non un intellettuale «puro» - un aggettivo che spesso si aggiunge a questa parola - perché tradirei il senso ultimo di quella ricerca, che non era mai solitaria e soprattutto non era mai avara. Segnare un progresso nella conoscenza, ma assai di più nella realtà e ancora di più nelle relazioni umane in termini di poteri, di diritti, di opportunità, per migliorarle progressivamente: questo era il fine. La sua speculazione incontrò Dio, lo ha ricordato Giacomo Caliendo. E ha detto poco, sono d'accordo, chi ha parlato di una sua conversione, perché senza alcuna paura Pietro Barcellona - e io mi chiedo a chi di noi basterebbe questo coraggio - disse che faceva i conti con l'ineludibile (nella vita di ciascuna persona) questione di Dio. E parlava di sé, ma leggeva il mondo e il peso che la religione ha nella sua storia e i mutamenti che questo ha indotto e ogni giorno induce nella vita di moltitudini umane e nella politica. Io lo voglio qui ringraziare. Ho mandato - direbbe lui - di ringraziarlo solo a nome di noi tutti ragazzi e ragazze degli anni chi più, chi meno, a seconda del coraggio di ciascuno di noi, ha insegnato a dubitare e a cercare, a non arrendersi alla banalità, a ciò che è scontato, al pressappochismo, all'ignoranza, alla mistificazione. E io vorrei, per le mie figlie, un maestro come lui. *(GAL)*. Signor Presidente, anche i senatori del nostro Gruppo si inchinano commossi alla memoria di Pietro Barcellona, avendo particolarmente apprezzato i profili che ne sono stati tracciati stamattina. Riprendendo dalla collega Finocchiaro questo bellissimo profilo dell'antidogmatismo di Pietro Barcellona, io, che non ho avuto il privilegio di essere suo studente, ma l'ho conosciuto quando ero già in quella fase di assistentino in carriera universitaria, ho sempre apprezzato di Pietro Barcellona l'antidogmatismo come altra faccia del miglior antiaccademismo della tradizione universitaria italiana. Pietro Barcellona significava una filosofia del diritto, sul tronco di una tradizione catanese di filosofia del diritto che Pietro Barcellona rispettava proprio perché non aveva nulla a che fare con la Catania del del crociano Bruno, del gentiliano Orazio Condorelli, del crocianissimo Vittorio Frosini. Ma le generazioni si succedono e mi è capitato di verificare, in morte di Pietro Barcellona, che, ben al di là dell'ancora giovanissima studentessa Anna Finocchiaro, Pietro Barcellona aveva incrociato addirittura la Catania di Pietrangelo Buttafuoco. C'era un ricordo di Pietrangelo Buttafuoco su «Il Foglio» a proposito di quell'incontro con l'ineludibile, che ad un certo punto l'uomo dell'antipositivismo giuridico, dell'anti-Kelsen, se volete dell'anti-Bobbio, dell'uso alternativo del diritto (per raccogliere una formula di

personaggi così discoli, così poco riconducibili a qualsiasi tradizione: appunto, Buttafuoco. E Buttafuoco rilevava, con la stessa eleganza di Giacomo Caliendo, l'incontro con Dio, l'incontro con un ratzingerismo del tutto inedito e inatteso. E in quell'occasione, in quella circostanza della vita, Pietro Barcellona aveva saputo raggiungere l'animo di Buttafuoco senza sperdere gli amici di sempre. Credo che il collega Tronti con maggior autorevolezza di me potrebbe ricostruire dall'interno di una coscienza quel processo. Ma è su tutta la figura e su tutta l'opera di Pietro Barcellona che i senatori del nostro Gruppo, in molta parte siciliani, si legano commossi e ringraziano i colleghi Caliendo e Finocchiaro di questa occasione. *(Applausi).* Signor Presidente, non voglio aggiungere altre parole a quelle già dette dai miei colleghi, ma semplicemente associarmi al ricordo del professor Barcellona, che personalmente conobbi, la cui figura sicuramente non si può relegare al solo ambito

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'annunziare il voto favorevole del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà alla Relazione

Mi pare sia emerso anche nella discussione in Aula, con lucida onestà, già dalla relazione introduttiva del presidente Azzollini, che il quadro economico e di finanza pubblica resta ancora oggi colmo di rischi e di incertezze. Sulla stessa linea, peraltro, il sottosegretario Baretta ha sottolineato che il documento che il Governo ha presentato è la testimonianza della complessità della situazione grave del nostro Paese. Non sappiamo dire se, come è stato detto ieri, il fondo sia già stato toccato e ci sia una vera ripresa o piuttosto ci siano incoraggiamenti che il Governo dà a sé stesso e al Parlamento rispetto alle prime azioni di questa prima fase di vita del Governo, ma dobbiamo avere chiaro l'Italia ha ancora una situazione economica e dei conti pubblici assolutamente incerta e fragile, con una serie di indicatori, che ieri in parte sono stati ricordati, assolutamente negativi. Mi riferisco al peggioramento dell'indebitamento, al calo dei consumi, al significativo crollo della fiscalità, che ci fa perdere un punto di PIL, a carico fondamentalmente del gettito IVA, alla marcata riduzione delle entrate delle accise energetiche al rischio concreto di mettere in ginocchio le entrate degli enti locali. I Comuni, non lo dimentichiamo, hanno difficoltà a chiudere i propri bilanci e ad approvare le loro effettive entrate. Vi è la necessità assoluta che il Governo si impegni con energia per impedire i ritardi che sono stati già ventilati nei pagamenti della pubblica amministrazione, rispetto ai quali Parlamento e Governo si sono impegnati in maniera significativa in questi ultimi mesi e in queste ultime settimane. A noi - ma non solo a noi - restano forti perplessità sulle coperture, come peraltro sottolineato dallo stesso presidente della Commissione bilancio, Azzollini. Pochi restano infatti gli interventi significativi che ci aspettavamo e ci aspettiamo ancora su tagli e sprechi. Restiamo lontani dalla concreta possibilità di una riorganizzazione reale di questo Paese, a partire dagli enti locali. Penso ancora alle Province, rispetto alle quali siamo tutti in attesa di sapere, con il rischio di vedere un comportamento da vecchie liturgie con le quali il rischio di pensare che il Governo abbia ancora un pizzico di coraggio in meno rispetto a quanto va fatto per riorganizzare dalle basi il sistema Paese. Restiamo inquieti quando le coperture vanno a toccare diritti, anche i più banali, che il cittadino aveva considerato un semplice esempio. Si riducono le detrazioni per le polizze vita, sulle quali molti cittadini avevano anche programmato una parte del loro incerto futuro. Agire sulle misure di detrazione o di deduzione fiscale per cercare coperture finanziarie è un errore grossolano perché si mina la fiducia dei risparmiatori e dei contribuenti onesti. Chi garantisce, ad esempio, che i contribuenti che ora vorranno accedere alle recenti misure del 50 per cento per le ristrutturazioni edilizie o a quelle del 65 per cento destinate all'efficientamento energetico degli edifici domani non si troveranno con la riduzione di queste agevolazioni, come si è fatto con le polizze vita? Abbiamo bisogno di certezze, delle cose più banali, che accompagnino il cittadino onesto nella sua difficile vita vita quotidiana. Nel decreto di fine agosto, inoltre, si creano o si implementano una serie di fondi per l'accesso alla casa, con il che si dà la sensazione di una sorta di novello statalismo con una presenza ingombrante dello Stato e con risultati economici e finanziari incerti a sostegno di ciò che noi vogliamo sia sostenuto, fondamentalmente se non esclusivamente, dal mercato. Nel decreto del fare si era prevista, e si è prevista, la impignorabilità della prima casa da parte di Equitalia, una disposizione che, al contrario, sembra di riflesso limitare, per gli indicatori di cui disponiamo, l'accesso al mutuo di molti soggetti. Abbiamo l'impressione che ancora si adottino misure estemporanee, mentre bisognerebbe adottare una seria politica per la casa, che costringa il sistema bancario ad essere al servizio del cittadino e dello sviluppo, perché questo Paese deve riprendere a produrre ricchezza. A proposito della casa, abbiamo l'esempio, già consolidato in altri Paesi dove la casa è, come da noi, un bene primario e dove si mira a preservare il valore dell'immobile. Possiamo riproporre tale esempio nel nostro Paese. Per consentire l'accesso ai mutui basterebbe consentire una detrazione totale degli interessi passivi sul mutuo. Si otterrebbe così un mercato libero, con un sistema creditizio vero e più forte, più aperto e più dinamico, con tassi di interesse più bassi,

questo sì, rilanciare il sistema del mercato immobiliare, perché il valore degli immobili si è polverizzato in questo momento nel nostro Paese, così come la fiducia dei cittadini. Non sono le tasse che fanno crollare questo mercato, ma la impossibilità di accesso al credito. Al contrario, non abbiamo letto alcuna misura per ridurre spese inutili, sprechi, privilegi, che pure ancora sono sotto gli occhi di ciascuno di noi. Né abbiamo letto misure di seria semplificazione per la vita dei cittadini e per le attività delle imprese.

si ripropongono di anno in anno, e i cicli, alla fine, sono fatti da curve che salgono e da curve che scendono. Ma non possiamo contare solo su questo. Abbiamo un disperato bisogno di fermare le partenze dei tanti giovani che se ne vanno e che lasciano il nostro Paese. Abbiamo un Mezzogiorno sempre più spopolato dal quale, nel 2050, spariranno milioni di *under* 44 tra denatalità, disoccupazione, nuove emigrazioni. Abbiamo una condizione di segregazione femminile, di impossibilità di accesso al lavoro. Abbiamo 20.000 laureati che dal Meridione si sono trasferiti all'estero negli ultimi anni. Abbiamo la necessità di confidare sul valore, l'impegno e la serietà di un Governo di grande coalizione al quale abbiamo chiesto, sin dal suo insediamento, che si impegnasse in un progetto di sviluppo radicale e complessivo del Paese, uno sviluppo che partisse dal Sud. Segni di questo tipo ancora non se ne vedono. Parliamo di documenti, come quello all'ordine del giorno del Senato, augurandoci che gli indicatori

Sia l'intervento del relatore che del Sottosegretario, ma soprattutto l'intervento di ieri del presidente Letta sul Vertice di San Pietroburgo rendono bene l'importanza politica di questo Documento, che ci fornisce indicazioni importanti e precise e che ci dice che, pure tra mille difficoltà e incertezze, oggi si registrano per l'Italia spiragli di ripresa. Non solo, ma, come ha detto bene il presidente Letta ieri, non siamo più sorvegliati speciali. Venendo ai contenuti, la Relazione contiene importanti interventi come il rifinanziamento della cassa integrazione guadagni per 500 milioni di euro; lavoratori cosiddetti licenziati individuali, che hanno lasciato il posto di lavoro prima della riforma pensionistica (qui si interviene a favore di circa 6.500 soggetti, un intervento sicuramente parziale, ma comunque un primo intervento); agevolazioni a favore delle categorie svantaggiate per l'accesso alla prima casa e interventi di sostegno al mercato immobiliare, e in particolare l'aiuto alle famiglie attraverso la Cassa depositi e prestiti; fondi per 200 milioni di euro per rendere più sostenibili gli oneri dei mutui e delle locazioni delle abitazioni attraverso diverse e importanti tipologie d'intervento; i pagamenti di parte dei debiti pregressi degli enti territoriali; la cancellazione per il 2013 della prima rata dell'IMU sull'abitazione principale e sui terreni e fabbricati agricoli; l'introduzione per il 2014, a regime, della *service tax*, che ci auguriamo alleggerisca il carico fiscale per le famiglie e, soprattutto, per le imprese. Attendiamo ora i provvedimenti attuativi e su questi avremo poi modo di discutere più a fondo e di affrontare nel merito i problemi. Come si vede, si tratta di provvedimenti importanti, ma in questo momento - ripeto - assumono un particolare significato politico che più volte è stato espresso in quest'Aula: l'assoluta necessità di non vanificare il lavoro fatto, l'assoluta necessità di non tornare indietro e far precipitare il Paese in una crisi drammatica, con conseguenze pesantissime sui mercati finanziari - ne abbiamo già avuto le avvisaglie - e sulla nostra credibilità internazionale, credibilità che stiamo, con grandi sacrifici di tutti, lentamente recuperando. I dati e le indicazioni contenute nel Documento, che mi auguro oggi approveremo, ci dicono che il Governo aveva fatto una valutazione giusta della situazione e che le misure introdotte erano corrette. Viviamo ancora in una situazione di forte rischio e ogni segnale di incertezza politica farebbe precipitare probabilmente la situazione. Colleghe e colleghi, oggi noi abbiamo una grande e pesante responsabilità: quella di trasmettere al Paese e alla comunità civile un segnale di fiducia e di stabilità politica. Abbiamo approvato provvedimenti importanti, altri li stiamo discutendo: penso alle importanti proposte per l'arte e il rilancio della cultura, al decreto delle semplificazioni, al disegno di legge per la razionalizzazione della spesa pubblica, al cosiddetto decreto del fare 2, alle importanti norme ambientali (per la cui urgenza abbiamo votato ieri), ai provvedimenti per i giovani e il lavoro, alle riforme fondamentali che sono già state impostate e che affronteremo Dobbiamo proseguire su questa strada per consolidare i pur tenui segnali di ripresa e per rispondere con responsabilità alle attese della popolazione. Mi auguro davvero che il Parlamento e tutte le forze politiche rispettino tale impegno.

insufficiente. Abbiamo cominciato questa legislatura con le Commissioni speciali, le quali hanno trattato prevalentemente questioni di natura economica e di funzionamento dello Stato, la prima questione trattata è stata quella dei debiti della pubblica amministrazione, centrale e periferica, nei confronti del sistema delle imprese.

secondo la Banca d'Italia erano 90, forse 100 miliardi di euro e secondo gli operatori, cioè le imprese e il sistema associativo democratico dei produttori, si arrivava a 130-140 miliardi di euro.

Non sappiamo come stia funzionando il sistema di pagamento. Noi speriamo funzioni benissimo;

Perché la pubblica amministrazione non ha pagato i propri debiti in modo puntuale, violando la legge? Era previsto che li pagasse in modo puntuale.

tutti coloro che hanno concretamente prodotto un buco che va, secondo le stime, dai 70 ai 140 miliardi di euro. Ecco la ragione per la quale noi non voteremo a favore di questa Relazione, che non è una ragione politica pregiudiziale, non è ideologica, ma è una ragione di merito: non c'è un atto di questo Governo che definisca una modalità chiara, certa, con la quale ritiene si debbano risolvere i problemi dell'economia e della finanza pubblica. Va a tentativi, produce iniziative scollegate dall'insieme, non c'è un ragionamento complessivo, se non una decisione: la spesa pubblica si deve fermare. Si deve fermare e non si deve correggere, non si deve revisionare, non si deve meglio orientare? Si deve solo fermare. Dall'altra parte, poi, abbiamo un PIL

gestire il declino inesorabile. Noi chiediamo che ci sia più coraggio che ci sia più coraggio per determinare un'inversione di tendenza. Noi vogliamo che ci sia un progetto di crescita,

nel sistema della speculazione finanziaria, a sentire i dati delle borse, si attestano, anche per l'Italia, nell'anno di crisi 2012 attorno al 7 Non c'è investimento privato che oggi abbia il coraggio di orientarsi alla produzione e all'impresa. Se non si muove l'investimento pubblico e non si combina e non si sollecita quello privato, noi non usciremo mai dalla crisi nella quale ci troviamo.

Per inquadrare il momento bisognerebbe però fare una piccola digressione e partire dal Governo Monti. Il ruolo che si è dato quel Governo probabilmente è stato l'inizio di una serie di gravi errori. Il Governo Monti ha puntato sul risanamento dei conti pubblici e ha completamente trascurato l'economia e la produzione. Ripianare i conti pubblici è una cosa relativamente semplice:

riparte. Il Governo Letta, sottosegretario Baretta, è un po' la prosecuzione, l'espressione della stessa maggioranza

non è che possono essere letti con la lente deformata in base al tasso di maggioranza che ognuno di noi ha nel sangue. Che cosa leggiamo nella Relazione? Sembra un mantra: il consolidamento fiscale. Se però non pensiamo alla ripresa dell'economia, che poi è l'unico elemento che lo sosterrebbe, mai più avremo consolidamento.

il dato ce lo dice - non riescono a mantenere quel tenore di vita che avevano in precedenza. I ceti medi stanno per scomparire perché non hanno nemmeno la garanzia e i supporti del *welfare*. La situazione è effettivamente preoccupante. Che cosa occorrerebbe in questa fase? Ci aspettavamo come minimo una riforma del sistema fiscale:

che metterli in moto sul mercato generando soltanto effetti positivi. Compensare tra imposte dirette e indirette: sappiamo che gli evasori non pagano le imposte. facciamo magari pagare in misura maggiore sui consumi, avremo anche un extragettito derivante dall'evasione che oggi sembra non si riesca a combattere.

Abbiamo chiesto che le risorse derivanti dall'efficientamento e dalla razionalizzazione della spesa pubblica vadano ad aumentare i fondi erariali a favore dei Comuni virtuosi. Lei ha risposto picche. Le ricordo che la collega Comaroli si è fatta approvare

Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, Scelta Civica voterà a favore della risoluzione che approva la Relazione del Governo. Siamo tutti consapevoli dei difficili equilibri della nostra finanza pubblica e della fatica di rispettare gli impegni assunti verso il nostro Paese e verso l'Unione europea, indispensabili per dare consistenza ai pur timidi segnali di ripresa. Se gli altri crescono e noi no dobbiamo ricercare nelle nostre lentezze, nella rigidità del nostro sistema, nelle nostre disfunzioni, soprattutto della pubblica amministrazione, la causa principale dei nostri mali. È per questo che la fine della recessione dipende soprattutto da noi. Per questo occorre stabilità politica e occorre investire le poche risorse disponibili a favore dell'unico fattore che davvero favorisca la crescita, vale a dire la riduzione della tassazione sulle imprese del costo del lavoro per creare un circolo virtuoso tra ricchezza, investimenti e occupazione. In un momento di crisi, all'uscita della crisi, occorrono segnali diversi rispetto a quelli dati dal decreto IMU, che è frutto di una mediazione politica e che potrà avere senso con le dovute correzioni e integrazioni solo se le priorità sul versante delle imprese e del lavoro verranno riaffermate, come ha garantito ieri il presidente Letta. Gli indirizzi di questa Relazione ribadiscono gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti dal Governo Monti e ribaditi dal Governo Letta. Per queste ragioni noi, richiamando qui integralmente qui integralmente quanto detto ieri della senatrice Lanzillotta, voteremo a favore, riservandoci di agire nel merito quando verrà trattato il decreto sull'IMU. Signor Presidente, colleghi leggendo la Relazione del Governo ho constatato l'avvicinamento del Governo al Movimento 5 Stelle. Però, dopo abbiamo visto che non si è avvicinato agli elettori, ma ha voluto agevolare probabilmente la stesura del prossimo spettacolo di Beppe Grillo. Spiego «Il complesso delle nuove misure avrà un impatto favorevole sull'economia e lascerà inalterato l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche riflettendosi unicamente sul fabbisogno finanziario e sul debito. Resta dunque confermato l'obiettivo di conseguire un saldo di indebitamento netto in rapporto al PIL entro la soglia del 3 per cento per l'anno 2013». Sì, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche potrebbe anche rimanere inalterato, ma quello dello Stato è in forte peggioramento. Con l'emissione di nuovo debito pubblico si riconosce un debito che per definizione non era conteggiato nel calderone, come ad esempio il debito commerciale delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese. C'era da scommetterci che il rapporto *deficit*-Pil debba stare a tutti i costi entro il 3 per cento. In realtà, la voragine nei conti pubblici non fa ben sperare. Nel 2012 il PIL, ai prezzi di mercato, è stato pari a 1.565,9 miliardi di euro correnti, con una riduzione dello 0,8 per cento rispetto all'anno precedente. In volume il PIL è diminuito del 2,4 per cento e per il 2013 nel DEF il PIL stimato è pari a 1.573,2 miliardi di euro. Ecco, alcune economisti stimano che il PIL per il 2013 sarà pari a 1.551 miliardi di euro. Che il PIL ce la mandi buona, altrimenti a fine 2013 avremo un rapporto *deficit*-PIL ben oltre il 3 per cento. Quello che si può dire con certezza è che l'Italia è l'unico Paese del G7 in cui il PIL non cresce, ma decresce. Secondo i dati diffusi pochi giorni fa dall'OCSE nel 2013 il PIL dell'Italia si attesterà a -1,8 per cento. Citando Citando ancora la Relazione del Governo: «La cosiddetta "crescita acquisita" fino a tutto il secondo trimestre del 2013 è pari a - 1,7

PIL. Ancora. Il Governo nella sua Relazione afferma: «Gli andamenti economici della prima metà del 2013 confermano la correttezza delle valutazioni effettuate dal Governo all'atto del suo insediamento e delle decisioni successivamente prese. Dopo il notevole consolidamento fiscale intrapreso nel 2012 e già programmato per il 2013 si è reso necessario affiancare alle politiche di riforma iniziative a sostegno dell'economia capaci di attenuare gli effetti recessivi Il calo della domanda, avvenuto nei primi mesi dell'anno, si è successivamente rivelato maggiore di quanto previsto, confermando ulteriormente l'importanza delle azioni intraprese. Queste ultime hanno contribuito a stabilizzare la situazione economica Come già emerso nei mesi scorsi, a causa della contrazione del PIL verificatasi nella prima parte dell'anno, e in particolar modo nel primo trimestre, la previsione di crescita annua contenuta nel DEF (...) dovrà essere rivista verso il basso». basso». Leggendo questi tre passaggi della relazione del Governo si intuisce l'ottimismo che accompagna il nostro *Premier*, mentre a noi non rimane che cogliere il modo schizofrenico e scellerato con cui chi ha la responsabilità politica si occupa della cosa pubblica. Con riferimento alle agevolazioni a favore delle categorie disagiate, per l'accesso alla prima casa e il sostegno al mercato immobiliare, facciamo attenzione, il Governo dice di intervenire prevedendo la messa a disposizione da parte della Cassa depositi e prestiti di una base di liquidità a favore delle banche - ci risiamo per l'erogazione di nuovi mutui per l'acquisto dell'abitazione principale, nonché l'acquisizione da parte della Cassa stessa di obbligazioni bancarie nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteche su immobili residenziali. Questo al fine di liberare l'attivo delle banche, che potranno così erogare nuovi mutui alle famiglie per l'acquisto di abitazioni principali. Speriamo che questa sia la volta buona, che le banche liberino il loro attivo bancario concedendo nuovi mutui alle famiglie. Speriamo che l'intervento non si trasformi nell'ennesimo regalo al sistema bancario: ne abbiamo già visti abbastanza. Quando le banche chiedono, con la minaccia di chiudere definitivamente i rubinetti del credito a famiglie e imprese, il Governo è solerte nel concedere aiuti, non ci pensa due volte. Quando a chiedere sono i piccoli imprenditori non ci sono le risorse; anzi, se si permettono di insistere li massacra ancora di più minacciando nuovi aumenti degli acconti acconti IRAP, IRES (c'è anche una clausola di salvaguardia in merito) e IMU. Dicevo che il peggio deve ancora arrivare; tra l'altro, dal 2015 avremo a che fare con un giochino infernale: la regola del debito o "*six-pack*", che stabilisce che gli Stati membri il cui debito superi il 60 per cento del PIL (quindi sicuramente noi) debbano ridurre tale rapporto ad un ritmo adeguato a convergere verso il valore di riferimento. Affinché la riduzione sia adeguata è necessario che la distanza del rapporto debito-PIL dalla soglia del 60 per cento si riduca al passo di un ventesimo all'anno, calcolato alla media dei tre anni antecedenti la valutazione. Il mancato rispetto del criterio del debito è valutato in base a tre condizioni e, se queste non vengono soddisfatte, si apre la procedura. Rispetto a quest'ultimo passaggio la Corte dei conti ha sottolineato che l'Italia, per garantirsi il pareggio di bilancio e il rispetto dei vincoli sul debito, deve avere un tasso di crescita nominale del PIL di un punto superiore a quello richiesto agli altri Paesi europei per i prossimi vent'anni. La Corte ha anche affermato che l'avanzo primario dell'Italia, sempre per rispettare i vincoli del debito, deve essere superiore a quello degli altri Paesi europei, anche nell'ipotesi che lo *spread* fra i vari Paesi europei e la Germania fosse azzerato. Sempre la Corte dei conti ha definito tale percorso un'ipotesi non realistica.

Questo non significa tuttavia che non sia stata una decisione assolutamente convinta quella che noi esprimiamo; convinta soprattutto perché nella Relazione al Parlamento predisposta dal Governo sono indicate le nuove misure che sono state adottate e che vanno tutte nel segno, più volte auspicato da noi e dalle altre forze di maggioranza, di intervenire su punti salienti della nostra economia. Innanzitutto, vi sono l'ulteriore finanziamento per il pagamento per il pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, il rifinanziamento della cassa integrazione guadagni, il sostegno ai lavoratori cosiddetti esodati (una piaga che bisognava risanare e che ancora non è interamente risanata, quindi va ulteriormente affrontata), le agevolazioni per l'accesso alla prima casa e il sostegno al mercato immobiliare; inoltre, vi è quella che consideriamo una misura estremamente positiva, ossia

sugli effetti sul bilancio dello Stato, con un aumento di 8 miliardi di euro. Infatti, quando si interviene per motivazioni assolutamente precise e giustificate, soprattutto con iniezioni di liquidità nel sistema che generano nuova ricchezza, allora anche il ricorso all'indebitamento può essere correttamente valutato, specialmente quando è parziale rispetto al cumulo degli interventi proposti. Questo deve essere però anche un campanello d'allarme, perché il ricorso all'indebitamento deve essere giustificato con provvedimenti assolutamente coerenti con la crescita, lo sviluppo e il superamento di alcune forti ingiustizie sociali frutto di

in particolare, il calo dei consumi, visto che abbiamo registrato nell'assestamento approvato due giorni fa un'ulteriore crescita di indebitamento causato dall'insussistenza di alcune voci delle entrate. Questo deve farci riflettere sull'eventuale possibilità di ulteriori aumenti di accise ed ulteriori aumenti di tassazione su settori che hanno segnato un calo dei consumi conseguente proprio ai precedenti aumenti.

negli anni passati e aumenti delle accise per coprire nuove sacche di precariato o nuove richieste del pubblico impiego sono aumenti che non ci possiamo permettere,

scolaretti che devono semplicemente ascoltare quello che dice qualche maestrina di turno). Noi dobbiamo essere consapevoli del nostro modo di agire e del fatto che possiamo passare a uno stato ancora più precario

la contrazione dei consumi alimenta un circolo negativo in tutta l'economia e non contribuisce certamente a creare le premesse per quella ripresa che tutti auspichiamo. il Gruppo del PD approva la Relazione presentata dal Governo in base alla normativa vigente di finanza pubblica. Questa occasione consente di svolgere una prima valutazione in merito agli andamenti macroeconomici della nostra economia e dei conti pubblici, mentre una discussione più articolata potremo svolgerla in occasione della presentazione da parte del Governo della Nota al DEF, prevista nei prossimi giorni. La Relazione si è resa necessaria in seguito all'approvazione del decreto-legge di fine agosto, che ha previsto un nuovo finanziamento degli ammortizzatori sociali, la cancellazione della prima rata dell'IMU, il riordino della tassazione sugli immobili, misure volte a sostegno delle famiglie sui mutui per la prima casa e gli affitti e un'ulteriore salvaguardia a favore dei lavoratori esodati. Si tratta di un complesso di misure volte ad arricchire il periodo di iniziative legislative che il Governo ha promosso in questi mesi per sostenere la ripresa economica e, al tempo stesso, salvaguardare le categorie di italiani che più hanno sofferto il dramma della crisi economica. Misure che in sede di conversione del decreto - come ha detto nel dibattito il senatore Fornaro - vanno sicuramente migliorate sotto il profilo dell'equità sociale. Misure, è bene ricordarlo, promosse entro confini di finanza pubblica estremamente ristretti dai vincoli di bilancio che resteranno tali nei prossimi tempi. Ma ora il quadro economico internazionale presenta prospettive migliori. Si evidenzia che le economie avanzate stanno finalmente uscendo dalla recessione e si iniziano a registrare i primi segni di ripresa. Anche il Centro Studi Confindustria ieri ha affermato ha affermato che si prevede una ripresa della crescita, seppur debole, già nel quarto trimestre del 2013. Dopo anni di grande difficoltà che hanno determinato nel 2013 dati ancora negativi sulle entrate, sulla crescita del debito, sull'aumento della disoccupazione, sono piccoli segnali positivi che non hanno ancora impatto sulle condizioni di vita dei cittadini, sulla tenuta dei livelli occupazionali ma che comunque non dobbiamo sprecare. E in questo quadro - lo diciamo al Governo - le misure delle prossime settimane saranno decisive. Noi abbiamo già indicato le priorità, che voglio qui brevemente riprendere: mettere in campo tutte le misure utili per completare rapidamente il pagamento alle imprese dei debiti della pubblica amministrazione, una misura che già oggi offre risultati importanti, ma che va attentamente monitorata rimuovendo tutti gli ostacoli burocratici; intraprendere con convinzione la strada della riduzione del peso fiscale sul lavoro e sulle imprese, come indicato anche dal documento congiunto sindacati- Confindustria; agevolare l'accesso al credito per le aziende; sostenere la domanda interna e i consumi. In parallelo, però, va affrontata con decisione la revisione della spesa, soprattutto per combattere con efficacia sprechi e inefficienze.

mentre sul piano istituzionale va attuato un robusto processo di semplificazione dei livelli istituzionali della struttura burocratica, come più volte indicato anche da provvedimenti del Governo oggi in discussione. Sarà altresì decisiva la capacità di utilizzare con più efficacia i Fondi europei, con una radicale discontinuità rispetto all'andamento fortemente deficitario del ciclo 2007-2013. Sono queste le direttrici fondamentali capaci di agganciare i primi deboli segnali di ripresa e di trasformarli, anche per l'Italia, in una possibile via di uscita dalla crisi. Non possiamo non rilevare come in questo quadro sia decisiva la tenuta politica dell'Esecutivo, condizione indispensabile per ogni ripresa economica. Le fibrillazioni di questi giorni hanno avuto preoccupanti ricadute sui mercati e sul costo del debito. È un prezzo che non possiamo far pagare ancora una volta ai nostri concittadini. raggiungimento della parità di bilancio e la conseguente fuoriuscita dalla procedura di *deficit* ci consentiranno nei prossimi mesi una limitata libertà di spesa, uno spazio di manovra che dobbiamo destinare integralmente al sostegno della produzione, degli investimenti e dell'occupazione. Per aggredire le basi istituzionali della crisi dovremmo anche accompagnare questi interventi con riforme efficaci capaci di affrontare il tema della riduzione dello *stock* del debito già nel 2014 per liberare risorse capaci di accorciare la distanza tra il nostro sistema produttivo e quello dei nostri competitori. però modo di sviluppare queste riflessioni e di supportarle con proposte concrete quando si discuterà la legge di stabilità, alla quale credo rinviamo una parte importante della nostra azione, al

Signor Presidente, colleghi, la questione che sottopongo alla vostra attenzione non ha, a mio parere, colore politico, né tanto meno rappresenta un problema riguardante solo il presente di tutti noi, ma è un tema che riguarda il benessere comune e il futuro del territorio del nostro Paese; territorio che da anni viene danneggiato da una politica fatta di provvedimenti normativi che spesso vanno in direzione opposta a quella auspicata da

rappresentanti dei cittadini, abbiamo il dovere civico e morale di fare in modo che le norme adottate da questo Parlamento provino la volontà concreta di salvaguardare l'ambiente e la salute delle persone. Ciò premesso, appare ora rilevante riassumere brevemente i due provvedimenti oggetto di contestazione, adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *pro tempore* dell'allora Governo Monti, i quali dimostrano l' esatto contrario di quanto detto in precedenza. Il primo provvedimento è il decreto ministeriale n. 22 del 14 febbraio 2013, recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), cui vengono stabiliti, tra l'altro, i criteri da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario cessino di essere qualificate come rifiuto. Il secondo provvedimento è il decreto ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2013, che modifica l'allegato X della parte quinta del codice ambientale, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario e che recepisce il decreto ministeriale n. che indica i criteri affinché determinate tipologie di combustibili solidi secondari cessino di essere qualificati come rifiuto e possano quindi essere riutilizzati. In sintesi, con i suddetti provvedimenti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *pro tempore* ha dimostrato la ferma volontà di proseguire in quella che appare la scorciatoia dell'incenerimento dei rifiuti nei cementifici, bruciando rifiuti solidi urbani per alimentare i forni di cottura del *clinker*, cioè la componente principale del cemento. È noto che l'Italia ha ricevuto numerose condanne da parte dell'Unione europea per le continue infrazioni della normativa in materia. Ciò che credo però debba interessare i colleghi, oltre alle infrazioni e alle condanne ricevute dal nostro Paese, è il fatto che si continui ad adottare provvedimenti normativi, come quello di cui discuto, che di fatto costituiscono un danno serio sotto il profilo della salute umana. L'utilizzo dei cementifici come inceneritori dà vita a polveri sottili, definite talvolta come «il nemico» oppure «il *killer* invisibile» dell'ambiente. Mi preme far presente che il decreto legislativo n. 152 del 2006 ha espressamente vietato l'immissione nell'atmosfera - si legge testualmente - di «qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa (...) che possa causare inquinamento atmosferico», costituendo un pericolo per la salute umana. Ebbene, il decreto legislativo n. 155 del 2010 individua, tra le principali attività produttive responsabili di emissioni in atmosfera, la produzione di cemento e i rifiuti utilizzati come combustibile. Quelli appena citati sono provvedimenti nazionali adottati per dare esecuzione a direttive comunitarie. Si ricorda che l'incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti sono disciplinati dalla direttiva 2000/76/CE. Detta direttiva comprende disposizioni speciali relative ai valori "limite di emissione" relativi ai forni per cemento che utilizzano i rifiuti come combustibile normale o addizionale. Il 24 maggio 2012 il Parlamento europeo ha approvato la relazione Gerbrandy su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, che invita la Commissione europea a razionalizzare la normativa in materia di rifiuti tenendo conto della gerarchia dei rifiuti e della necessità di ridurre quelli residui fino a raggiungere l'obiettivo rifiuti zero. Per questo, il testo chiede alla Commissione di presentare proposte, entro il 2014, allo scopo di introdurre gradualmente un divieto generale dello smaltimento in discarica a livello europeo e di abolire progressivamente, entro la fine di questo decennio, l'incenerimento dei rifiuti riciclabili e compostabili. Alla luce dei suindicati provvedimenti normativi e degli intendimenti programmatici delle istituzioni comunitarie, non è comprensibile come sia stato possibile adottare due decreti ministeriali che di fatto vanno in direzione diametralmente opposta a quella dettata dal legislatore comunitario e nazionale. Ma, ad avvalorare quanto sin qui osservato, è d'obbligo evidenziare anche l'*iter* seguito dall'allora Ministro, con il quale sono stati adottati i due decreti di cui si discute. Antecedentemente all'adozione del citato decreto ministeriale, l'allora Ministro dell'ambiente aveva presentato al Parlamento, per il parere, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'utilizzo di combustibili solidi secondari da bruciare nei cementifici. Il medesimo schema di decreto del Presidente della Repubblica aveva però ottenuto parere negativo da parte della Camera, e quindi il Ministro ha ben pensato di avocare a sé il potere di legiferare, sottraendo al Parlamento il potere che gli è riconosciuto dalla Costituzione. Questo è un atto grave, che merita di essere censurato. In conclusione, la scelta dell'incenerimento dei rifiuti nei cementifici non può e non deve essere condivisa, in quanto, in primo luogo, essa è certamente contraria alla normativa comunitaria e nazionale. In secondo luogo, essa espone l'Italia ad ulteriori condanne da parte della comunità europea. In terzo luogo, continuare a bruciare rifiuti è uno spreco di risorse e costituisce un costo altissimo in termini ambientali e di salute dei cittadini. È dunque necessario, in conclusione, che il Governo si impegni ad abrogare il decreto ministeriale n. 22 del 14 febbraio 2013, attuativo, per i combustibili

possano cessare di essere qualificate come un rifiuto e diventare un combustibile alternativo, e non ne sia quindi conseguentemente consentita la libera circolazione al di fuori delle singole Regioni. 2) ad abrogare il decreto ministeriale 20 marzo 2013 recante "Modifica dell'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS)", che recepisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di CSS cessano di essere qualificate come rifiuto, di cui al suddetto decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22. Colleghi, fino ad oggi abbiamo assistito a continue dimostrazioni di incapacità della classe politica di proporre soluzioni in linea con quei principi di sostenibilità ambientale che da decenni l'Europa ci chiede. del disegno di legge Atto Senato n. 941, meglio conosciuto come il decreto salva-Ilva, questa Camera dichiara di essere costretta, per motivi di urgenza, ad approvarlo nonostante fosse dichiaratamente e palesemente contro ogni regola di buon senso: ora, oggi, abbiamo invece la possibilità di approvare un provvedimento tutti insieme, per dimostrare che non siamo recidivi nel fare sempre le scelte sbagliate. Ve lo chiedo come collega, come parlamentare e come cittadina.

solidi secondari (CSS) da rifiuti a sottoprodotti consente ai cementifici di utilizzare nella produzione di cemento i CSS come combustibili,

marciano bene e in linea con l'Europa, con percentuali di raccolta differenziata molto elevate e quindi con comportamenti virtuosi, vi sia un'altra parte del Paese che continua a lavorare a lavorare in piena emergenza. Anche questo provvedimento è frutto, ancora una volta, di questa filosofia: una filosofia per la quale, dopo anni e anni, si continuano a emettere provvedimenti che sono fatti sull'onda dell'emergenza. E sull'onda dell'emergenza vengono adottati provvedimenti che sono - ahimè! - certamente non coerenti con la strategia europea e che noi riteniamo

questo non lo affermiamo noi, ma lo affermava già il ministro dell'ambiente Clini in varie interviste, in cui sponsorizzava l'utilizzo dei combustibili

Tra l'altro, vorrei qui ricordare che queste affermazioni nonché questi decreti hanno un aspetto molto discutibile da ogni punto di vista, che i cementifici, di fatto, possano utilizzare il CSS non tiene conto del fatto che gli stessi sono già delle industrie insalubri di classe prima, che hanno limiti di legge da rispettare,

di emissione adeguati a quello che viene bruciato, cioè veri e propri rifiuti.

il cementificio è «un impianto altamente inquinante, con e senza l'uso di rifiuti come combustibile, e produce almeno il triplo di CO2 rispetto a un inceneritore classico». classico». Quindi, dal punto di vista ambientale e dell'impatto sulla salute, si tratta di un'operazione non solo discutibile, ma molto di più. Inoltre, vorrei ricordare che i limiti di emissione di inquinanti per questi impianti

di diossine è proporzionale alla quantità di rifiuti bruciati", i microinquinanti emessi dai cementifici potrebbero essere "maggiori rispetto a quelli degli inceneritori" i dati che il Ministero dell'ambiente aveva all'epoca portato a suffragio della bontà di questo decreto sono dei dati che, già di per sé, ci dicono che

I cementifici, in questo modo, già di per sé hanno molti problemi. Bruciando i rifiuti (perché di questo stiamo parlando), generano un impatto ambientale molto ampio, non confinabile soltanto al nanoparticolato. Tra l'altro, vorrei ricordare che il nanoparticolato può viaggiare per distanze molto ampie sospinto dal vento. Il nanoparticolato è la frontiera ultima della ricerca e della scienza in ambito medico, tanto che quella parte della ricerca spesso sovvenzionata dagli stessi colossi energivori dell'incenerimento dei rifiuti tende a minimizzare gli effetti derivanti dalle micropolveri emesse dalla dalla combustione, anche ad altissime temperature. Ed è questo uno dei problemi maggiori, proprio dal punto di vista dell'impatto sanitario. Tra l'altro, francamente noi riteniamo assolutamente sospetta la fretta con cui un Governo dimissionario aveva varato il decreto propedeutico al decreto del Presidente della Repubblica.

a ignorare e disattendere le disposizioni europee sul recupero della materia secondo le quali sono gli interventi finalizzati alla raccolta differenziata quelli prioritari, e non l'uso di metodologie distruttive che ignorano, tra l'altro, altre direttive. Tutto questo peraltro è costato all'Italia la condanna

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, il problema dei rifiuti rappresenta indubbiamente una grande emergenza ambientale del nostro Paese. Più propriamente dovremmo considerarlo una patologia cronica, in quanto emergenza richiama una temporaneità che non corrisponde al lungo perdurare nel tempo di una situazione, come nel caso del problema dei rifiuti. attestano questa realtà e io ne cito alcune. Quattro Regioni (Campania, Sicilia, Lazio e Calabria) sono al collasso; quasi un terzo della popolazione nazionale con grandi aree urbane come Roma, Napoli e Palermo sono coinvolte. discariche, a fine febbraio 2012 abbiamo ricevuto una comunicazione di messa in mora da parte della Commissione europea per la presenza sul territorio nazionale di 102 discariche non conformi alla direttiva 1999/31/CE che imponeva di adottare entro il luglio 2009 misure di chiusura o di adeguamento delle stesse. Nonostante ciò procediamo con intollerabile lentezza nel regolarizzare tali anomalie e in realtà, se non vogliamo mentire a noi stessi, la situazione sul territorio è ben peggiore di quanto non risulti dai dati ufficiali: centinaia e centinaia di discariche pubbliche (non parlo di quelle illegali, altro dolente capitolo) esaurite e abbandonate sono disseminate ovunque, di fatto ignorate, senza progetti e senza risorse per la bonifica, e rappresentano una macchia indelebile per il territorio. procedure di infrazione, il numero e la portata delle procedure aperte a nostro carico per il mancato rispetto delle normative comunitarie ci ha tristemente caratterizzato come paese fuorilegge. Nel 2010 la Corte europea di giustizia ci condanna per la mancata creazione di una rete integrata di gestione dei rifiuti urbani nella Regione Campania e nuovamente veniamo deferiti alla stessa Corte nel giugno di quest'anno per i ritardi nell'attuazione dei programmi concordati. La Commissione europea ha proposto di sanzionarci con una somma forfetaria di circa 30 milioni di euro per il passato e una penalità di mora, qualora l'inadempimento perdurasse, pari a 250.000 euro al giorno. Le ecoballe, una montagna di rifiuti di otto milioni di tonnellate, sono imballate e stoccate nei vari siti in Campania in attesa di smaltimento. Non è un caso se tra i Paesi dell'Unione europea siamo agli ultimi posti nella classifica per l'efficienza nella gestione dei rifiuti. una situazione che chiama in causa la credibilità stessa del sistema politico-istituzionale che, in materia di rifiuti, ha assunto troppo spesso come regole di comportamento il sottrarsi alle proprie responsabilità e l'acquiescenza alle cattive abitudini, come fa oggi chi, vagheggiando 1'utopia futura del rifiuto zero, sfugge al compito delle risposte ai problemi frutto di un passato di disattenzioni, superficialità e scelte sbagliate. Ancora, nel 2010 in Italia veniva conferito in discarica poco meno del 50 per cento dei rifiuti, mentre la media dell'Unione europea è del 37 per cento (la Germania è all'1

con l'unica eccezione del 2011-2012 dovuta esclusivamente alla forte contrazione dei consumi. Nel 2010 abbiamo prodotto 32,5 milioni di tonnellate di rifiuti, oggi sfioriamo i 30 milioni Ma le più accreditate previsioni indicano una ripresa del *trend* di crescita dei rifiuti nei prossimi anni, e ciò rende veramente inderogabile la necessità di ridurre i conferimenti in discarica che rappresentano la vera anomalia

nonché uno spreco enorme di energia (il valore economico corrispondente al potere calorifico di rifiuti urbani smaltiti in discarica è stimato in oltre un miliardo di euro). Vista la dimensione del problema e poiché l'entrata a regime di una politica che si sviluppi attorno a prevenzione-riduzione, riuso e riciclo richiederà tempi lunghi, occorre gestire una fase transitoria che non può prescindere dal ricorso, pur limitato, al recupero energetico attraverso termovalorizzazione. È altrettanto evidente che la realizzazione di nuovi impianti risulta particolarmente complessa e controversa; per questo si è fatta strada l'ipotesi di utilizzare impianti già esistenti e in esercizio come i cementifici dotati di forni per la cottura del *clinker*, componente essenziale del cemento, forni alimentati da combustibili fossili che possono essere efficacemente sostituiti da combustibile proveniente da rifiuti. È il caso del CSS, prodotto derivante dal trattamento di alcuni rifiuti, del quale prima il decreto legislativo n. 152 del 2006 e successivamente il decreto ministeriale n. 22 del 14 febbraio 2013 fissano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo in impianti industriali quali cementifici. In Europa questa è una strada già ampiamente praticata: in Olanda e in Germania il CSS rappresenta rispettivamente l'83 e il 62 per cento del combustibile utilizzato nei cementifici.

utilizzo di impianti già esistenti; sostituzione di un combustibile fossile che dobbiamo importare, con un combustibile alternativo prodotto da noi con evidenti vantaggi in termini di bolletta energetica (valutati da Nomisma in 368 milioni di euro annui). A fronte di queste opportunità, sono stati sollevati timori sul fatto che l'utilizzo di CSS possa compromettere i progetti di raccolta differenziata, ma occorre tenere conto che le stesse caratteristiche merceologiche del CSS necessitano a monte di una selezione dei rifiuti. Inoltre, esso viene prodotto utilizzando quasi esclusivamente rifiuto non riciclabile che altrimenti verrebbe smaltito in discarica. Le preoccupazioni emerse riguardo alle eventuali negative ricadute sull'ambiente e sulla salute delle emissioni conseguenti all'utilizzo del CSS nei cementifici sono le più serie e non vanno sottovalutate a patto che non siano pretesto di ostilità pregiudiziali e strumento per la ricerca di facili consensi. Quindi, si rendono certamente necessari approfondimenti e valutazioni attente e prudenti. Comunque, il quadro normativo e le risultanze dei più qualificati studi scientifici sono incoraggianti in tal senso. A livello europeo, l'uso di CSS nei cementifici è previsto come una delle migliori tecniche disponibili; in Italia il suo utilizzo è limitato alle cementerie con capacità produttiva superiore a 500 tonnellate al giorno e pertanto soggette ad AIA e alla normativa sul coincenerimento dei rifiuti, in linea con le analoghe direttive europee. Per quanto riguarda le emissioni dei cementifici rispetto agli inceneritori, anche in questo caso gli studi scientifici segnalano che le emissioni sono generalmente inferiori rispetto a quelle prodotte da combustibili Gli unici limiti per i quali la norma prevede valori più elevati sono quelli degli ossidi di azoto nonché delle pm 10, ma per entrambi sono stati verificati effetti migliorativi con l'utilizzo del CSS rispetto ai combustibili fossili. Per le diossine, in particolare, le alte temperature dei forni (oltre mille gradi) garantiscono la distruzione e l'ossidazione di tutte le molecole inquinanti di natura organica. Ciò non vuol dire che l'adozione di tale sistema ci renda immuni da ogni impatto o ricaduta negativa, ma poiché è innegabile che la gestione dei rifiuti in Italia comporti ancora oggi costi inaccettabili a carico della natura e delle persone, sarebbe da stolti rinunciare aprioristicamente a ricercare e praticare soluzioni in grado di attenuare, se non di eliminare, tali problemi. In conclusione, l'utilizzo del CSS non può essere lo strumento per trasformare i cementifici in inceneritori, ma per garantire ad essi 1'utilizzo di un combustibile alternativo a quello fossile per contribuire ad assolvere agli impegni europei in materia ambientale ed offrire soluzioni concrete a specifici problemi del nostro Paese. Un moderno ed integrato ciclo di gestione dei rifiuti deve necessariamente coniugare le ragioni della fattibilità tecnica e praticabilità economica con quelle della tutela dell'ambiente e ancor più della salute delle persone. I troppi casi di negligenze, omissioni e drammatici errori che hanno determinato tragedie ambientali ed umane hanno seminato sfiducia e avversione verso la politica e le istituzioni. La risposta non può essere certo 1'immobilismo, che rappresenterebbe, come è accaduto fino ad oggi, il danno più grave per il nostro Paese, ma scelte rigorose trasparenti e capaci di rassicurare, come quelle che chiediamo al Governo con questa mozione. Signor Presidente, onorevoli senatori, la Lega Nord ha da sempre affrontato le questioni ambientali come temi che partono dal basso, ossia dalla popolazione, e ha sempre indicato le proprie posizioni che possono essere prese come modello e costituire tendenza ed elemento portante per l'azione dell'uomo. Senz'altro non condividiamo l'azione del Governo Monti che, ad inizio anno, da una parte ha sospeso l'Atto del Governo n. 529 sull'utilizzo del CSS nei cementifìci, perché non condiviso dal Parlamento, e dall'altra, con un atto di forza, lo ha sostanzialmente sostituito, in realtà provocando effetti analoghi, prima con il decreto ministeriale n. 22 del 2013 e poi con quello del 20 marzo 2013.

evidenziano una posizione di freno relativo alle infrastrutture e sono contrarie *a priori* alla pratica di bruciare i rifiuti, indipendentemente dal fatto che tale pratica sia utilizzata per il recupero di energia termica o elettrica negli inceneritori o nei termovalorizzatori e indipendentemente dal fatto che tale pratica possa essere effettuata a seguito di un processo di gestione del ciclo dei rifiuti che comunque preveda la raccolta differenziata e il recupero delle materie prime potenzialmente recuperabili. A nostro avviso, la debolezza dei due testi consiste principalmente nel fatto che non è vero che la raccolta differenziata rappresenta la soluzione al problema e non lo potrà essere forse per sempre. Lo diciamo per esperienza fatta sul campo in qualità di ex amministratori locali che hanno contribuito a sviluppare forme di gestione eccellenti al Nord, con punte di differenziazione del 70 e 80 per cento, *compost* compreso. Inoltre, tali mozioni creano allarmismo in ordine all'inquinamento, senza tenere conto che i cementifìci sono impianti altamente inquinanti anche se bruciano gasolio o carbone e che l'utilizzo di combustibile in luogo del carbone comporta anzi un abbassamento delle emissioni. Senza contare che già oggi, cari colleghi, i cementifici (e sono pagati per farlo) sono autorizzati a bruciare rifiuti di ogni genere come farine animali, pneumatici, il CDR, che oserei definire il papà del CSS, ma anche il semplice CSS che già oggi esiste sul mercato. seconda considerazione è che resta indiscutibile che il Paese deve stabilire una linea chiara di riferimento per quanto riguarda la produzione di energia e la riduzione delle emissioni, sia quelle climalteranti, sia quelle dannose per la salute della popolazione. Ma a fianco di tali problematiche si pongono quelle, in certi casi drammatiche, dello smaltimento dei rifiuti, le quali si presentano come cattive pratiche, tipiche e quasi esclusive del nostro Paese, di diffuse zone del Sud (in Sicilia, in Calabria e a Napoli, dove pesano anche economicamente le multe inflitte dall'Europa per le reiterate infrazioni), ma anche del centro (Roma su tutte con la discarica di Malagrotta, che ritornerà nei prossimi giorni a rappresentare un'emergenza, una vergognosa emergenza). In tale ambito spicca un'azione catastrofista, talvolta alimentata dai *media*, che ha demonizzato alcuni modelli di smaltimento dei rifiuti, come l'incenerimento e la termovalorizzazione. Si tratta di un'azione origine del lassismo, che ha paradossalmente giustificato l'inerzia di molti amministratori incapaci del Centro-Sud, responsabili di diffuse pratiche di mala gestione del ciclo rifiuti. Azioni catastrofiste che, per taluni soggetti, hanno anche rappresentato il punto di forza e poi il successo della propria campagna elettorale anche nel Centro-Nord. La Lega Nord ha condiviso da sempre una posizione a favore di una riduzione dei rifiuti. I Comuni e le Province amministrate dalla Lega Nord, nei distinti ruoli, hanno da sempre proposto ed attuato forme di gestione dei rifiuti che hanno raggiunto un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Tuttavia, siamo convinti che dopo la riduzione, la differenziazione, la selezione e il recupero di materia da rifiuto, occorre pensare anche alla possibilità di produrre energia attraverso il trattamento dei rifiuti residuo. Questo deve avvenire in modo tale da fornire un'ulteriore opportunità a tutta la comunità. Pensiamo ai termovalorizzatori, al teleriscaldamento, alla possibilità di utilizzare rifiuti per la produzione di energia termica, invece che materie fossili peraltro non infinite. Le politiche ambientali sono legate, da una parte, al sistema di informazione, educazione e sensibilizzazione del cittadino verso tematiche ambientali e, dall'altra, al controllo delle emissioni, con particolare riferimento all'abbassamento delle emissioni degli inquinanti atmosferici da parte di impianti industriali, mezzi di trasporto, impianti termici ed energetici. Anche la scuola può giocare un ruolo importante sulla formazione dei giovani alle politiche ambientali. Ci sono esempi importanti. Consentitemi di menzionare un progetto che si sta attuando ormai da una decina di anni nel mio Comune di Calolziocorte, dove fino a pochi mesi fa sono stato sindaco. Ogni anno tutte le classi (una ventina) della scuola media inferiore vengono messe in sana competizione tra loro a chi raccoglie più carta. Ad ogni studente delle prime tre, le quali arrivano a raccogliere ciascuna fino a 20 tonnellate di carta, viene dato un buono acquisto del valore di 20, 10 e 5 euro. Inoltre, alla scuola quale premio generale viene data una dotazione informatica. È questo un piccolo esempio virtuoso, un progetto tra scuola, Comune e società pubblica che gestisce la raccolta dei rifiuti. terza e ultima considerazione è che l'Italia non può restare indietro rispetto ai nostri *partner* europei e deve comunque governare la produzione di combustibili solidi secondari (CSS), e in particolare il distinto CSS-combustibili di maggiore e certificata qualità. qualità. Ribadiamo che l'obiettivo deve essere quello di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, ivi incluse le emissioni di gas climalteranti, all'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile a scopi energetici della biomassa contenuta nei rifiuti, ad un più elevato livello di recupero dei rifiuti stessi. L'incenerimento dei rifiuti per la produzione di energia termica comporta senz'altro una riduzione degli oneri ambientali ed economici legati allo smaltimento di rifiuti in discarica e con l'uso controllato del CSS nei cementifici esistenti che sottolineo continueranno a rimanere tali e non verranno trasformati in inceneritori - forse e finalmente si potrà dire la parola fine ai problemi vergognosi del Centro-Sud, con discariche spesso abusive e tanti commissari inutili e dispendiosi. Con la nostra mozione chiediamo al Governo di impegnarsi, prima di qualsiasi azione diretta, a disciplinare l'utilizzo del CSS nei cementifici, a promuovere comunque un approfondito dibattito sulla materia da parte delle Commissioni parlamentari competenti, fornendo un quadro aggiornato sull'attuale utilizzo del CSS e del CSS-Combustibile nei cementifici, sia in Italia, disaggregato per Regioni, sia all'estero, che possa analizzare la questione attraverso apposite audizioni dei rappresentanti delle Regioni e dei soggetti economici coinvolti ed approfonditi esami di studi scientifici Gli approfondimenti dovranno in particolare fare riferimento: alle emissioni di sostanze inquinanti e alle possibili conseguenze sul piano ambientale, sanitario e sociale, anche a seguito ad eventuali malfunzionamenti o errori di gestione (in ogni caso, i limiti imposti dall'AIA per le emissioni dovranno essere analoghi a quelli previsti per gli impianti dedicati alla termovalorizzazione); alle conseguenze del traffico indotto relativo al trasporto del CSS e alle ripercussioni del traffico indotto sulle realtà territoriali soprattutto, alle restrizioni che occorre individuare circa la circolazione in altre Regioni del CSS proveniente da rifiuti urbani, garantendo comunque il criterio di prossimità e che gli impianti di trasformazione dei rifiuti urbani in CSS siano comunque situati all'interno di ciascuna Regione dove vengono prodotti i rifiuti (in sostanza, i rifiuti urbani siciliani, calabresi, campani o laziali devono essere trattati nelle stesse Regioni); al rispetto rigoroso della gerarchia di gestione dei rifiuti prevista dalle direttive comunitarie nella catena della produzione sia del CSS-Combustibile, sia del CSS normale, allo scopo di evitare

in relazione ai progetti in essere per l'utilizzo di combustibili alternativi da parte dei cementifici; infine, al rafforzamento, con ogni strumento a disposizione e su tutto il territorio nazionale, del sistema dei controlli sia sulle emissioni inquinanti dei cementifici mediante una rete di monitoraggio ambientale sia sul processo di gestione dei CSS utilizzati in tali impianti sia sul trasporto e la tracciabilità del CSS, onde scongiurare fenomeni malavitosi, e sia sul rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti ai fini della produzione del CSS. *(Applausi

Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando si bruciano i rifiuti - e il CSS è di fatto un rifiuto - si formano delle sostanze: diossine, metalli pesanti e particelle. Le diossine, una grande famiglia di 200 composti, sono veramente molto pericolose e si concentrano nel nostro corpo per quel processo chiamato biomagnificazione. Se fosse vero quello che avete detto che a 1000 gradi le diossine spariscono dovreste spiegare quello che è successo a Mantova. In questa città avevamo un bellissimo inceneritore che ha bruciato tutta la diossina di Seveso. La concentrazione qualitativa e quantitativa della diossina di Seveso è esattamente quella che c'è a Mantova, per cui se a 1.000 gradi sparisce perché dovrebbe esserci? Lavori sperimentali dell'Università della Louisiana del 2006 e oggi studiosi canadesi, confermano che quando si brucia diossina, durante la fase di raffreddamento dei fumi questa si riforma. Quindi, non è vero che gli inceneritori fanno sparire la diossina.

e una volta nel sangue creano un problema di tromboembolie. Studi dell'Università di Milano dimostrano che chi vive vicino alle autostrade dove ci sono tante particelle muore di più di *ictus* e di tromboembolie polmonari. Inoltre, queste sostanze passano nel sangue e quando la donna è incinta le si trovano nei bambini malformati. Che le nanoparticelle siano pericolose lo sa benissimo il presidente Formigoni, che con due delibere regionali del 2008 del 2009 ha invitato i cittadini a non accendere le stufe a legna nel periodo autunnale in pianura perché producono le nanoparticelle. Purtroppo io sono un medico, sono un patologo e per giunta di Mantova. Ho eseguito 2.500 autopsie e potrei farvi vedere le nanoparticelle non solo nei feti malformati, ma anche nei cani, nei gatti, i quali non fumano, come dice il commissario dell'Ilva. Potrei dire molte cose, ma i quattro minuti a mia disposizione stanno terminando. Vorrei ricordare che le ceneri vengono messe nel cemento e qui il nostro intonaco libera piombo e mercurio, che poi noi ci respiriamo. È già stato detto che sono contro la Comunità europea. Occorre ricordare, comunque, che già nel 1960 i medici sapevano che l'asbesto provocava il mesotelioma e ci abbiamo messo trent'anni per fare una legge. Ora sono quindici anni che i medici sanno queste cose. Quanto tempo dobbiamo aspettare? Quanti morti dovremo piangere?

*(M5S)*. Signor Presidente, io innanzitutto sono anche un medico, e volevo evidenziare che la combustione dei rifiuti in parziale sostituzione dei combustibili fossili è una pratica che rende immediatamente disponibili per l'incenerimento dei rifiuti, con una procedura estremamente semplificata, i 59 cementifici localizzati sul territorio nazionale, che si sommerebbero ai già tanti inceneritori disponibili: l'Italia è infatti al terzo posto in Europa per numero di inceneritori operativi. Non è di rifiuti inceneriti che abbiamo bisogno né degli inquinanti e delle ceneri tossiche prodotte da tale pratica. Ci si domanda allora perché non ci si ispiri al principio di precauzione, a partire dalla COM (2001) 31 della Commissione europea, che dovrebbe essere adottata nei casi in cui vi siano sospetti di conseguenze negative sulla salute dei bambini, ma non evidenze scientifiche consolidate. In questa occasione mi voglio rivolgere a tutti i colleghi medici presenti in quest'Aula, a qualsiasi Gruppo parlamentare essi appartengano. Credo che ogni medico debba avere a cuore la salute dei suoi pazienti e dei cittadini tutti. Come medici siamo a conoscenza dei rapporti tra ambiente e salute: non è un caso che ne stiamo discutendo in 12a Commissione. Continuiamo ad immettere nell'ecosfera sostanze di tutti i tipi, in gran parte tossiche, che stanno provocando cambiamenti repentini, con conseguenze - come abbiamo sentito - che colpiscono sia adulti che bambini e (cosa preoccupante) anche molte donne in gravidanza. Ritengo che come medici dobbiamo prima indignarci e subito dopo combattere contro queste pratiche scellerate. Le malattie croniche (come il diabete di tipo 2, l'obesità infantile, le malattie neurovegetative e le malattie autoimmuni) sono in aumento esponenziale in tutto il mondo, e sono state messe in relazione con i cambiamenti ambientali, causati prevalentemente dall'immissione in ecosfera di inquinanti da parte di attività industriali che si basano su processi di combustione ad alte temperature. Sentiamo spesso che il problema della sanità è l'infiltrazione decisionale della politica: come medici senatori, facciamo in modo che la sanità da noi rappresentata nelle istituzioni legislative sia libera dagli errori e orrori della classe politica. *(Applausi Facciamo capire ai nostri colleghi senatori che noi siamo qui per difendere la salute, non solo di coloro che ci hanno votato o sostenuto, ma di tutti gli indifesi di fronte alle nostre scelte sbagliate, anche in buona fede.

di ridurre la produzione di rifiuti, di favorire le buone pratiche; soprattutto, vorrei che i rifiuti rappresentassero una fonte di lavoro, di economia e un bene comune e non solo un oggetto di profitto e un bene per le *lobby* produttrici di combustibili solidi secondari e di cemento.

facciamo qualche appunto tecnico. La direttiva 2008/98/CE, che è quella grazie alla quale siamo arrivati a fare questa bella definizione di combustibile solido secondario,

poi recuperi, eventualmente bruciando, e poi, se proprio non ce la fai, butti via il rifiuto. Le buone esperienze italiane ci dicono che si può arrivare a buttar via il 4 per cento, seguendo correttamente la gerarchia. Peraltro, andando più avanti, questa direttiva dice: se proprio non riesci a rispettare la gerarchia, perché tecnicamente non ce la fai o perché economicamente non è praticabile o per questioni di protezione ambientale, puoi puoi anche fare altro. Ma tutte queste ostruzioni non ci sono, perché in Italia ci sono buone pratiche in base alle quali questi tre problemi non sono tali, e lo diventano solo se qualcuno ritiene di voler fare qualcos'altro con questi rifiuti. Il concetto è che con questa direttiva ti viene anche detto che in certe condizioni puoi promuovere e non degradare da rifiuto a materia prima-seconda: è una promozione. Vorrei allora sapere - e non solo io - con che testa uno dice che,

bruciamo il rifiuto nei cementifici, che sono dei forni, in quanto producono calore, non hanno nessun tipo di recupero di altro genere. Ricordiamo che il recupero puramente termico è ancora meno efficiente del recupero in un inceneritore, e noi già non siamo d'accordo con gli inceneritori, figurarsi se siamo d'accordo con questa pratica di bruciare questi benedetti CSS nei cementifici. Concludo dicendo un'altra cosa. Qui ho sentito un aborto dal punto di vista termodinamico. Qualcuno infatti è assurdo prendere questi oggetti ed utilizzarli in altro modo, perché potremmo recuperare tutta l'energia termica che c'è dentro: risparmiamo sulla bolletta energetica se bruciamo queste sostanze.

ho preparato un breve testo per spiegare questa materia che è abbastanza complessa e si presta anche a facili strumentalizzazioni. Procederò in sintesi e poi esprimerò il parere sulle vari mozioni. CSS (combustibili solidi secondari) si colloca nel complesso degli interventi di politica ambientale, energetica e industriale di cui l'Italia necessita al fine di assolvere agli impegni europei e internazionali in materia ambientale ed energetica. In tal senso la produzione e l'utilizzo del CSS-combustibile offre un significativo potenziale. Il crescente prezzo del petrolio e di altri combustibili primari (ad esempio, il *coke* di petrolio e il carbone fossile), sintomo di un'incipiente scarsità aggravata da un generale contesto di crisi economica, rende urgente la ricerca di fonti energetiche alternative. L'Italia è uno dei Paesi industrializzati maggiormente dipendenti da importazioni dall'estero di fonti di energia, e ciò determina cronici squilibri della bilancia dei pagamenti. Considerazioni di carattere strategico impongono, inoltre, di garantire la massima diversificazione del *mix* energetico, la riduzione della dipendenza dalle fonti fossili e una maggiore sicurezza e stabilità degli approvvigionamenti. Considerando lo scenario, è quindi necessario promuovere non soltanto lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma anche l'utilizzo di combustibili alternativi,

la cui valorizzazione in determinati comparti industriali (cementifici, centrali termoelettriche) consente di trasformare un problema in una risorsa per un settore produttivo e per la collettività. Alcune tipologie di combustibili solidi secondari presentano qualità merceologiche tali da giustificare, sotto profili normativi, il loro inquadramento come un autentico prodotto combustibile. L'utilizzo di combustibili alternativi, con particolar riguardo ai combustibili solidi secondari prodotti da rifiuti, è anche particolarmente indicato sotto profili di politica industriale. Il crescente utilizzo di combustibili basati sulla biomassa vergine, ad esempio, desta anche preoccupazioni sotto il profilo economico, in quanto provoca distorsioni nel mercato dei prodotti alimentari (cereali, mais ed altro) e di alcune importanti produzioni industriali nazionali (carta, mobili e quant'altro) contribuendo a ridurre la dipendenza da combustibili importati e a favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/CE. In aggiunta alle sfide derivanti dalle tematiche sopra delineate, l'Italia si trova a dover inoltre affrontare alcuni problemi prettamente nazionali legati alla gestione dei rifiuti. La quantità di rifiuti costituisce un problema ambientale e territoriale comune a tutti i Paesi industrializzati, ma con connotati ma con connotati più gravi per l'Italia e, in particolare, per alcune aree del nostro Paese che fanno ancora ampio ricorso allo smaltimento in discariche, di cui molte fra l'altro in via di esaurimento. La prassi dello smaltimento in discarica rappresenta non soltanto un potenziale rischio ambientale, ma anche un enorme spreco di risorse materiali ed energetiche quali sono i materiali che possono essere ottenuti, previa effettuazioni di recupero, dai rifiuti. Sebbene l'esportazione dei rifiuti praticata da alcune Regioni italiane verso altri Stati membri contribuisca a risolvere, nell'immediato, le gravi emergenze in corso, si tratta di pratica insostenibile nel lungo periodo sia in considerazione dei costi ambientali ed economici del trasporto e del trattamento sia in ragione delle perdite economiche nette derivanti dal mancato sfruttamento dei materiali e delle risorse energetiche contenute nei rifiuti spediti, a titolo oneroso, all'estero. Sotto questo profilo, occorre urgentemente pianificare e realizzare in Italia alternative valide, mirando a conseguire l'autosufficienza a livello nazionale. Nel contesto energetico, ambientale e industriale sopra descritto, il decreto ministeriale n. 22 del 2013 offre un importante contributo alla soluzione delle evidenziate problematiche. Coerentemente con i dettami dell'articolo 184-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, stabilisce regole affinché la produzione e l'utilizzo di determinate tipologie di combustibile solido secondario avvengano nel più rigoroso rispetto degli *standard* di tutela dell'ambiente e della salute umana. 22 del 2013 ha istituito una specifica disciplina giuridica per regolamentare la produzione e l'utilizzo del combustibile solido secondario in alcuni impianti industriali prescelti che, per le garanzie fornite in campo ambientale e tecnico, sono particolarmente idonei a questo fine. L'utilizzo di combustibili alternativi in cementifici è pratica comune e diffusa in ambito europeo, in particolare in Paesi membri con elevate percentuali di raccolta differenziata ed in testa alla classifica europea dei Paesi virtuosi per la gestione dei rifiuti, dai quali spesso diciamo di voler prendere esempio. Appare pertanto semplicistico e comunque non corretto tecnicamente identificarlo con l'incenerimento, trattandosi di processi industriali assolutamente distinti e con notevoli specificità. Inoltre, si ricorda che l'utilizzo di combustibili solidi secondari in cementifici è riconosciuto, attraverso una recentissima decisione normativa (decisione della Commissione europea del 26 marzo 2013), a livello europeo come

in Europa cementerie che hanno raggiunto un livello pari al 100 per cento, sostituendo integralmente i combustibili fossili con i combustibili alternativi. Le cementerie italiane potrebbero realizzare percentuali di sostituzione simili o superiori a quelle degli altri Paesi, in tutta sicurezza. Dall'attuale 10 per cento di sostituzione termica, le cementerie italiane potrebbero tecnologicamente essere in grado già oggi di arrivare a livelli del 50 per cento, valore almeno confrontabile a quello del tasso di sostituzione raggiunto in Germania.

combustibile, a sua volta ottenuto da un processo di recupero di materia. Il decreto ministeriale n. 22 del 2013 è volto a far sì che la produzione e l'utilizzo di determinate tipologie di combustibile solido secondario avvengano nel più rigoroso rispetto degli *standard* di tutela dell'ambiente e della salute umana.

Il nostro è un documento che considero molto più equilibrato e costruttivo rispetto a quelli presentati da altre forze politiche e sui quali esprimo voto contrario, anche perché non condivido i toni allarmistici che sono stati usati in quest'Aula. Il tema affrontato è certamente delicato, ma va comunque

non fare nulla, per poi lasciare il problema alle discariche di Roma e trovarci nella situazione attuale non sia assolutamente un buon comportamento. Ritengo che il problema vada affrontato e, secondo noi, la produzione di combustibile solido secondario diventa a questo punto necessaria per evitare ulteriori conferimenti in discarica. Inoltre, le emissioni conseguenti ai trattamenti nei cementifici offrono più garanzie rispetto a quelle di un inceneritore, perché i limiti sulle emissioni imposti ai cementifici sono più restrittivi rispetto a quelli imposti agli impianti di incenerimento, le temperature sono più alte e i tempi sono più lunghi e dunque ciò garantisce un più completo incenerimento dei rifiuti e quindi emissioni «più pulite». In buona sostanza, un cementificio dà quindi maggiori garanzie rispetto a un inceneritore. Quindi, a nostro parere, va riconfermata la linea adottata dal precedente Governo, ma prevedendo cautele molto specifiche, un monitoraggio costante e precise precauzioni, che sono tutte contenute ed elencate in maniera rigorosa e precisa all'interno del documento che io stesso ho sottoscritto e che ci dà, come già detto, tutte le garanzie necessarie. Inoltre, l'utilizzo di combustibile solido nei cementifici dà una boccata d'ossigeno a un settore che sta vivendo, per lo stato dell'edilizia, una pesante crisi. Anche in Provincia di Trento, si è deciso che il cementificio di Sarche di Calarino possa utilizzare i fanghi residui dei depuratori per l'alimentazione energetica degli stessi impianti: ciò permetterà di evitare l'uso di *pet coke*, attualmente utilizzato, che è un combustibile molto più sporco. In tal modo si eviteranno trasporti inutili, si recupereranno fanghi residui e soprattutto avremo emissioni più pulite. Questa operazione peraltro consentirà al cementificio, che non diventa assolutamente un inceneritore (perché gli inceneritori trattano tutt'altro tipo di rifiuti) di ridurre i costi energetici e quindi garantire gli attuali livelli produttivi e occupazionali.

Prima di proseguire nelle dichiarazioni di voto, vorrei dare una comunicazione all'Assemblea. il Presidente della Repubblica mi ha comunicato di avere nominato, con decreto in data odierna, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il professor Giuliano Amato giudice della Corte costituzionale.

Signor Presidente, senatrici e senatori, non vi nascondiamo una forte preoccupazione. Abbiamo assistito, non solo in questa discussione, ma anche nei giorni scorsi, ad un quadro di assoluta inadeguatezza rispetto alla dimensione del problema. Sul piano ambientale e delle condizioni di vita e di salute nel nostro Paese, dobbiamo sapere che non è allarmismo quello che sto e che stiamo facendo nella discussione di oggi: abbiamo intere, importanti e strategiche aree del nostro Paese a rischio di crac ambientale.

sul livello di irrespirabilità dell'aria o circa l'impossibilità di bere l'acqua persino dagli acquedotti, perché con percentuali di inquinamento e di veleni tali da determinare la morte per gli esseri umani e per gli esseri viventi; abbiamo aree strategiche del nostro Paese già entrate in questo cono d'ombra.

io dico: attenzione, fermiamoci, perché le motivazioni presentate dal Governo,

di portare a bruciare milioni di tonnellate di qualcosa di cui spesso in Italia (non stiamo parlando di chissà quale altro Paese) nessuno è in grado di dire la la composizione e gli effetti sulle emissioni. Questa è la situazione del nostro Paese, questa è la situazione che c'è a Roma e nella Provincia di Roma; questa è la situazione che c'è nell'area della valle del Sacco, epicentro Colleferro, con un cementificio, con un termovalorizzatore, con incidenti che si sono già determinati. Quindi non stiamo parlando di quello che potrà accadere, ma stiamo parlando di qualcosa che è alle soglie del crac ambientale. Abbiamo già pagato milioni di euro per le infrazioni che ovviamente l'Europa ci sanziona. allora rovesciare questa piramide. È evidente che il discorso è diverso quando si affronta l'esempio di alcuni Paesi virtuosi, europei e non, in cui alla fine della filiera c'è un prodotto assolutamente individuabile.

Credo che in questo senso si debba fare attenzione, perché, se noi vogliamo muoverci nel costruire un circuito virtuoso, bisogna capire prima cosa mettere alla testa della piramide;

di vita all'interno di quei territori vasti. Ecco, cerchiamo di saperci fermare prima, cambiando però il taglio delle nostre iniziative,

Grazie

indipendentemente che si tratti di inceneritori, termovalorizzatori o cementifici, a prescindere dalla possibilità della riduzione delle emissioni e dalle garanzie che occorre assicurare ai cittadini circa l'adozione delle migliori tecniche sostenibili e l'effettuazione di severi controlli e indipendentemente dal fatto che tale pratica possa essere effettuata a seguito di un processo di gestione del ciclo dei rifiuti che comunque preveda la raccolta differenziata e il recupero delle materie potenzialmente recuperabili. C'è da dire che tutte e tre le mozioni, anche quella presentata dalla maggioranza, non fanno distinzione tra l'utilizzo del CSS,

rifiuti, previa AIA regionale: bruciano farine animali, pneumatici fuori uso e rifiuti in genere e sono pagati per farlo, e bruciano anche CSS che già esiste sul mercato. In Italia, Germania, Austria, Finlandia e Regno Unito l'utilizzo industriale del CSS e di prodotti analoghi a fini energetici costituisce una pratica industriale consolidata. L'inserimento di limiti a garanzia della qualità del CSS e per il controllo delle emissioni operato dal decreto ministeriale non modifica in realtà la situazione attuale, anzi potrebbe introdurre elementi di qualità che però vorremmo verificare attraverso un'opportuna discussione, che chiediamo nel dispositivo della nostra mozione. La nostra mozione si distingue dalle altre anche per alcuni paletti che intende inserire nel dibattito sulla possibilità di bruciare CSS o CSS-Combustibile nei cementifici, riconoscendo che si tratta di una situazione complessa su cui è necessario fare chiarezza e che richiede un approfondito esame da parte del Governo da subito ed anche del Parlamento, che deve coinvolgere il mondo economico e gli enti territoriali interessati.

Pertanto, c'è senz'altro un incremento del traffico indotto dal trasporto dei materiali, che aumenta dell'80 per cento e presuppone una diversa organizzazione del trasporto, per non creare impatti insostenibili dalle realtà territoriali locali. Tali aspetti devono essere considerati nell'ambito delle autorizzazioni degli impianti da parte delle Regioni. Inoltre, c'è da tenere conto del fatto che, come evidenziato nella nostra mozione,

privilegiando il criterio della prossimità ai fini del recupero e dello smaltimento, che permette alle amministrazioni di ridurre i costi aggiuntivi di trasporto ed evita ai cittadini di prestare il proprio territorio per smaltire i rifiuti di altri territori; l'eccellenza raggiunta dai comuni del

dove vengono prodotti i rifiuti. La trasformazione dei rifiuti in CSS non deve diventare la scusa per permettere il trasferimento dei rifiuti urbani al di fuori del territorio regionale. I cittadini devono essere poi adeguatamente informati a monte, e non a valle, di decisioni importanti come quelle prese dal decreto; e devono essere informati su ciò che succede nel proprio territorio e sui progetti che le Regioni e i singoli cementifici intendono mettere in atto per l'utilizzo di combustibili alternativi e di quelli di provenienza fossile. Purtroppo, in tema di controlli esistono marcate differenze fra le varie realtà territoriali del Paese. Quindi, una rete di controlli carenti, spesso con il compiacimento delle amministrazioni locali, può rendere il sistema labile, permettendo l'inserimento della criminalità organizzata nel ciclo della gestione dei rifiuti. Occorre pertanto rafforzare il sistema dei controlli su tutto il territorio nazionale sia attraverso una rete di monitoraggio ambientale delle emissioni inquinanti dei cementifici sia attraverso verifiche e accertamenti sul processo di formazione e gestione dei CSS utilizzati in tali impianti. La possibilità di bruciare CSS o CSS Combustibile nei cementifici si presenta pertanto come una situazione molto complessa, della quale le comunità dei territori che vivono intorno ai cementifici sono molto preoccupate. Pertanto, noi richiediamo un approfondito esame da parte del Governo e del Parlamento, che deve coinvolgere anche il mondo economico e gli enti territoriali interessati. La nostra mozione attesta comunque un approccio pragmatico

Grazie

Grazie perché noi non ci accontentiamo che il Governo valuti l'opportunità di fare questi approfondimenti. Come Gruppo della Lega Nord, riteniamo che questi approfondimenti debbano essere fatti a monte.

le mozioni in votazione nascono in risposta al decreto emanato lo scorso febbraio dall'allora ministro dell'ambiente, Corrado Clini, per utilizzare i per utilizzare i rifiuti solidi urbani per alimentare i forni di cottura del *clinker*, cioè la componente principale del cemento. Tale provvedimento è stato emanato in attuazione e coerentemente con le disposizioni europee in materia. È una soluzione che si rifà al principio dell'*end of waste*, ossia alla cessazione della qualifica di rifiuto prevista dall'articolo 6 della direttiva europea sui rifiuti del 2008, scopo di alleggerire il problema dello smaltimento dell'immondizia, anche scippandolo al circuito della malavita organizzata. La sostituzione dei combustibili tradizionali con i combustibili alternativi è fortemente avversata da alcuni ambientalisti, per i quali la combustione di rifiuti nei cementifici comporta una variazione della tipologia emissiva di quegli impianti, in particolare di diossine e metalli pesanti. È bene chiarire che non si tratta delle famose ecoballe, tanto meno di rifiuti presi tali e quali dalle strade, ma di combustibili ottenuti da un trattamento industriale complesso e regolamentato da specifiche norme di legge. L'impiego dei CSS nei cementifici è pratica largamente diffusa in tutto il mondo avanzato, con in testa l'Europa, che l'ha persino dichiarata una delle migliori tecniche disponibili. Così in Olanda, Germania, Francia e Austria (e non credo che questi siano Paesi che non hanno a cuore dei loro cittadini), tanto per fare degli esempi, i CSS costituiscono gran parte del combustibile utilizzato nei forni da cemento. Quelli citati sono peraltro tutti Paesi dove la raccolta differenziata è a livelli molto più elevati che in Italia (in Germania, ad esempio, è al 50 per cento). Ciò dimostra come riciclo e recupero non siano in contraddizione. In Germania, Olanda e Austria bruciano nei cementifici rifiuti di Napoli trasformati in CSS. In Italia, la domanda di CSS è a tutt'oggi bloccata per la complessità degli *iter* burocratici a causa del mancato consenso sociale: quando si parla di bruciare, scatta immediata la rivolta. Si tratta di 6 milioni di tonnellate di rifiuti che potrebbero essere assorbite dall'industria: oggi, invece, siamo fermi a 600.000 tonnellate. Perché in Italia siamo fermi all'8 per cento, nonostante gli immensi problemi di gestione dei rifiuti che hanno i nostri Comuni? Evidentemente molti nel nostro Paese hanno interesse a continuare nel ricorso alle discariche, sprezzanti delle varie infrazioni che la UE ha comminato all'Italia in materia, o nella costruzione di nuovi inceneritori, incuranti delle inevitabili proteste della popolazione. Nel frattempo i nostri concorrenti europei utilizzano i rifiuti spediti a caro prezzo del nostro Paese e li trasformano in CSS per impiegarli nei loro processi industriali. Quanto alla formazione delle diossine, questa dipende dalla presenza di cloro e delle temperature di combustione; in realtà nei cementifici la presenza di cloro nei forni è minima, sia per questioni di processo sia per rispetto della qualità del prodotto finale. Dunque, non solo non c'è nessun danno per la salute, ma la produzione e l'utilizzo dei CSS contribuisce a minimizzare il ricorso alle discariche e ridurrebbe la tassa sullo smaltimento dei rifiuti di circa il 14 per cento, secondo alcune stime.

La stessa Legambiente ammette che bruciare CSS nei cementifici non peggiora le emissioni inquinanti e, anzi, impone limiti di legge più restrittivi e, quindi, l'utilizzo di migliori tecnologie di abbattimento. Come sostiene Stefano Ciafani, vice presidente di Legambiente, «bruciare CSS nei cementifici li rende più controllati. Li obbliga a monitorare alcuni inquinanti - come le diossine - che la legge non impone di controllare quando bruciano altre schifezze come il *petcoke»* (carbone derivato dalla distillazione dal petrolio) «o il polverino di carbone, ben peggiore del CSS». Queste sono le cose che bruciano adesso nei nostri cementifici. Secondo l'ambientalista, quindi, «a parità di risultati, bruciare CSS in un cementificio è meglio che in un inceneritore sotto il profilo delle emissioni di CO2, fermo restando che i cementifici emissioni ne producono a prescindere, inquinano di per sé e dal punto di vista della salute sono comunque un problema». Questa è la citazione. e del Movimento 5 Stelle sono basate su ingiustificati allarmismi, nel presupposto - errato - che pratiche industriali applicate ordinariamente in altri Paesi siano nocive per la salute. Pertanto, annuncio il voto contrario del nostro Gruppo su questo. La mozione firmata anche dagli esponenti in Commissione ambiente di Scelta Civica impegna il Governo a trovare il giusto equilibrio fra difesa dell'ambiente, produzione industriale e smaltimento dei rifiuti. Dà, a nostro avviso, il giusto peso alla protezione della salute delle popolazioni che si trovano a vivere nei pressi dei cementifici, perché condiziona lo smaltimento dei CSS nei condiziona lo smaltimento dei CSS nei cementifici al rispetto di precisi parametri e controlli ambientali. Nello stesso tempo, va nella direzione di ridurre il vantaggio competitivo che oggi hanno i produttori di cemento stranieri per il fatto di poter utilizzare i CSS, potrebbe alleviare i costi dei Comuni (e quindi dei cittadini) per lo smaltimento dei rifiuti. Ancora una volta, come già per la questione dell'Ilva di Taranto, è necessario trovare un compromesso alto fra sviluppo economico, rispetto dell'ambiente e difesa della salute pubblica. *(Applausi

ha ragione il collega Arrigoni a dire che noi siamo contrari all'incenerimento. Ma questa non è una posizione ideologica: noi siamo contrari all'incenerimento dopo almeno sette anni di studi e audizioni, prima come cittadini semplici e adesso anche come istituzione. Abbiamo audito sul CSS i medici per l'ambiente. I dati riportati non sono ideologici: sono dati certi e accurati di studi scientifici. Quindi - mi dispiace di avere più tempo dei miei colleghi medici che avevano molto da dire e l'hanno dovuto fare in fretta - dobbiamo rilevare che con l'incenerimento dei rifiuti abbiamo chiaramente una materia eterogenea e difficilmente controllabile; abbiamo un incremento

ci hanno spiegato che con l'aumento del calore le particelle PM10 (che sono quelle dell'inquinamento) si disgregano, perdono massa e diventano fino a 1.000 o anche 2.000 volte più piccole; quando si raffreddano, a differenza delle diossine ,che tendono a riaggregarsi, per mancanza di massa non hanno la capacità di riaggregarsi e quindi restano polveri sottili, che arrivano nei feti. Ho visto le fotografie che il collega Gaetti ha prodotto nei suoi studi, e vi invito ad effettuare una ricerca, perché questa non è ideologia. Invito tutti voi, che avete una responsabilità enorme, ad approfondire

più volte siamo stati ripresi dall'Unione europea. Anche per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti, è stata citata l'ultima relazione europea del maggio 2012, là dove si afferma che la gerarchia dei rifiuti va assolutamente

già pronto nel cassetto! Anche questo è stato evidenziato, ma io vi voglio far ragionare. Perché questa forzatura, questa fretta, questo nuovo

Commissione della Camera (una decisione assunta con coscienza: bisogna leggere le motivazioni del rifiuto)?

la legge italiana prevede che basta fare un'accurata selezione manuale. Questo significa trasformare un rifiuto in un sottoprodotto? A mio parere, non è così. Infatti, è stato anche detto che non abbiamo impianti tali per trattare il rifiuto e trasformarlo in CSS,

Di Battista, ma non sono Di Battista). Potremo dire all'Europa che il CSS non è un rifiuto. Quindi, vai! Brucialo!

che «l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana». Questo non ci sta. Quindi, a mio parere, il CSS non può rientrare

urbano commisto a rifiuti speciali e bruciato in impianti impattanti, di categoria 1, che sono nocivi per la salute. Ma noi non diciamo che bruciare olio o carbone nei cementifici non sia un problema: è un problema. Ma bruciare i rifiuti è un problema maggiore, non solo perché il prodotto che si brucia è eterogeneo e difficilmente controllabile, si brucia una materia che si deve recuperare. Il problema della termodinamica, cui ha fatto riferimento il mio collega Martelli, è un dato reale.

infinito che possiamo consumare senza limiti. Questo è un mondo circolare: quello che prendiamo dobbiamo reimmetterlo nel circolo. È un mondo circolare.

Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, il nostro Gruppo voterà convintamente a favore della mozione presentata dalla maggioranza, a prima firma del senatore Morgoni. Essa propone un articolato insieme di indicazioni relative al potenziale utilizzo del combustibile solido secondario in alcune specifiche tipologie di impianti industriali: nella fattispecie i cementifici. Il documento si pone quale espressione di una prima fase di indirizzo orientata a rispondere con iniziative concrete, vorrei dire «del fare», a problematiche complesse in materia ambientale e di tutela della salute che richiedono urgenti interventi ad integrazione delle politiche sino ad oggi attivate, alla luce del crescente aumento della produzione dei rifiuti e della ricerca di nuove soluzioni, alla luce, inoltre, della necessità di fornire, in tutte le fasi di attuazione, chiare indicazioni alle comunità locali più prossime agli impianti. Data la vastità della materia è possibile soffermarsi solo su qualche punto. Il primo punto è il seguente. In particolare, la mozione richiede al Governo una serie di azioni che, se lette in maniera isolata, possono sembrare scontate ma per le quali, al contrario, si richiede un'analisi d'insieme, finalizzata ad evidenziarne la significatività metodologica e la potenzialità di sistema. Mi spiego. Ciò che nel complesso la mozione richiede con forza e immediatezza è un'attività di comparazione con esperienze in essere, di attenta analisi e di approfondimento tecnico-scientifico sugli effetti di ciascuna azione, senza che preconcetti, conclusioni affrettate carenza di verifiche dichiarino *a priori* la percorribilità o la non percorribilità di una soluzione. Il secondo punto che mi pare opportuno evidenziare è il seguente. Va ricordato che il riutilizzo ai fini energetici e produttivi del combustile solido secondario è già stato oggetto di apposita disciplina, in in particolare - come previsto dal decreto ministeriale n. 22 del 2013 - per quanto concerne le attività di controllo. esiti di approfondimenti scientifici sperimentali hanno consentito di rilevare un miglioramento dell'impatto emissivo delle combustioni praticate nei cementifici allorquando si è fatto ricorso al CSS in co-combustione. Tuttavia, si pongono quesiti cui rispondere in dettaglio in merito al connubio tecnologia - salute umana - e ambiente. In terzo luogo, ferma restando, dunque, una costante attività di ricerca tecnica che consenta di aggiornare le condizioni tecnologiche ed operative alle quali attenersi scrupolosamente per permettere l'utilizzo del CSS negli impianti industriali, si propongono al Governo iniziative collegate strettamente con il concetto di trasparenza nell'applicazione di processi industriali. Proprio al fine di far convivere il pragmatismo delle iniziative con la tutela della salute dei cittadini e la compatibilità con l'ambiente, si prefigura un sistema nel quale l'utilizzo del combustibile solido secondario sia oggetto di monitoraggio e informazione costante. Oltre alla previsione di norme specifiche per il completo rispetto delle disposizioni comunitarie e alla costituzione di appositi organismi di controllo, si pone in evidenza

in tal modo si avvia un sistema di confronto chiaro e dinamico con il territorio ove gli impianti sono collocati. Tra l'altro, va detto che questo schema di controllo degli effluenti e di monitoraggio e di comunicazione delle condizioni di esercizio può essere garantito con efficaci e affidabili sistemi di rilevazione degli indicatori, generali e puntuali, a fronte di costi ridotti. È evidente, poi, come un sistema di autorizzazioni all'esercizio, strutturato sulla base di elementi di chiarezza e attrezzato per fornire continue informazioni, rappresenta uno strumento di maggiore garanzia per il buon esito degli investimenti troppo spesso soggetti, nel nostro Paese, a continue incertezze vorrei dire incertezze fino all'ultimo bullone, con una battuta - con la dannosissima conseguenza di scoraggiare gli investitori. Il quarto punto da evidenziare è il Si tratta, dunque, di condividere un metodo che successivamente porti alla costruzione di un modello attuativo di maggiore garanzia rispetto alle politiche sin qui seguite. Va da sé che un tale passo richiede altresì di ricercare con costanza ed obiettività gli strumenti che dimostreranno il maggior grado di adeguatezza a tutte le problematiche sottese. La mozione fornisce in tal senso un insieme di indicazioni metodologiche molto puntuali (ben dodici punti) che richiedono una forte garanzia di serietà dell'approccio. Tra questi vi è l'impegno di aggiornare, ad esito dell'*iter* suggerito, la normativa di settore. In quinto luogo, si reputa opportuno richiamare la confortante esperienza - anch'essa citata dalla mozione e in altri interventi - di altre Nazioni europee, in alcune delle quali il riutilizzo dei rifiuti nei rifiuti nei cementifici è una pratica largamente diffusa, collaudata, ritenuta vantaggiosa per l'ambiente se raffrontata con l'uso di combustibili fossili e con pratiche di elevata compatibilità. Le tecnologie applicate hanno consentito di far riconoscere a livello europeo la combustione dei CSS come la miglior pratica disponibile con tassi di sostituzione termica dei combustibili fossili

In sesto luogo, nel complesso le azioni di analisi, informazione e monitoraggio sono dunque chieste al Governo da subito, affinché la pratica dell'utilizzo dei combustibili solidi secondari diventi eventualmente efficacemente operativa e vorrei dire serenamente applicabile anche nel nostro Paese, inserendosi tra le buone pratiche volte a garantire una soluzione a lungo termine nel trattamento dei rifiuti o di una porzione di essi attraverso, sia chiaro, la predisposizione di linee guida specifiche cui attenersi con scrupolo. Molti altri punti potrebbero essere evidenziati a supporto dei contenuti della mozione. Ciò che maggiormente merita un'ultima sottolineatura è la necessità di implementare - va ribadito - una nuova impostazione metodologica rispetto al problema di cui si sta trattando. In le scelte di azione o di non-azione non dovrebbero essere frutto di sentimenti ideologici, ma richiedere approfondimenti senza pregiudizi rivolti ad una totale trasparenza dei risultati scientifici acquisiti a vantaggio dei cittadini, delle imprese e per il futuro stesso del nostro Paese. *(PD)*. Signor Presidente, senatrici e senatori, il problema dei rifiuti e del loro smaltimento è uno di quei temi la cui risoluzione sarà strategica per il futuro del nostro ambiente ed anche, penso, per la svolta La situazione è complessa ed io invito tutti ad affrontare con l'ottimismo della buona volontà alcuni blocchi ideologici impegnandoci a mettere in campo tutte le energie derivanti dalle nostre preoccupazioni per intervenire là dove la norma ce lo permette per migliorare e focalizzare la nostra attenzione soprattutto sui temi della salvaguardia della salute e della tutela dell'ambiente. La discussione in Aula è stata approfondita e puntuale. Registro i quattro punti che su questo problema ci vedono preoccupati e coinvolti. La produzione del rifiuto è ancora troppo elevata ed è caratterizzata da una crescita che è in controtendenza rispetto ai dati dell'Unione europea a 27. a 27. Il fenomeno dello smaltimento illegale dei rifiuti industriali, ma direi anche della gestione delle discariche e della gestione della raccolta dei rifiuti è ancora troppo oggetto di attenzione delle ecomafie e del malaffare. Il Paese deve fare delle scelte illuminate, finalizzate alla riduzione del rifiuto, allo smaltimento/utilizzo del medesimo e questo deve essere fatto al meglio, alla lotta al malaffare che attorno al sistema dei rifiuti lavora e si sviluppa. Il rispetto per l'ambiente, l'aria, l'acqua e il suolo e, soprattutto, della salute dei cittadini con proposte e strumenti tali da dare risposte valide alle legittime preoccupazioni dei cittadini per la loro salute e anche degli operatori che sul mercato devono operare. Nonostante un movimento di forte sensibilizzazione e di coinvolgimento delle famiglie, dei comparti produttivi e del commercio, la produzione del rifiuto non tende a calare. Risparmio all'Assemblea, che è attenta ed informata, i dati relativi alla produzione del rifiuto del nostro Paese in rapporto a quelli europei. Ma mentre in Europa nell'ultimo quinquennio il consolidamento dell'attuazione delle politiche e delle normative comunitarie volte alla riduzione dei rifiuti destinati alla discarica e, in particolare, dei rifiuti biodegradabili, ha dato buon frutto, in quanto si è registrata una riduzione importante nella produzione dei medesimi, il nostro Paese, in controtendenza, vede (sono dati ISPRA) nel 2010 un aumento dell'1,1 rispetto al 2009, con una produzione di poco meno di 32,5 milioni di tonnellate di rifiuti urbani. Quello che ci preoccupa di più, però, è che, sempre sulla base dei dati ISPRA, più del 50 per cento di questi rifiuti continua ad essere smaltito in discarica. Noi abbiamo quindi bisogno di una politica che parta da subito con una visione lungimirante e complessiva su questa materia, che vada a definire soluzioni integrate, al raggiungimento degli obiettivi europei (in quanto abbiamo visto che hanno dimostrato la loro efficacia sui dati di *report*) e soprattutto in linea con quella che è definita la gerarchia delle attività, cioè la prevenzione, il trattamento per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero (tuttavia, quando parliamo di recupero dobbiamo anche sottintendere che è previsto il recupero energetico; questo non lo possiamo dimenticare) la loro destinazione tombale attraverso il loro smaltimento in discarica o nell'inceneritore. Se vogliamo prevenire l'utilizzo delle discariche e degli inceneritori per i conseguenti rischi di inquinamento ambientale e sulla salute

una politica forte sul riciclo e sulla prevenzione. Quindi, a questo punto, non possiamo dimenticare che il recupero ai fini della produzione di energia è una delle vie attuabili.

provengo da una Provincia della quale sono stata anche amministratrice, la Provincia di Cuneo, che all'interno del ciclo integrato dei rifiuti, gestito interamente dal pubblico, utilizza fino a ieri il CDR-Q e oggi il CSS all'interno di un cementificio. Avere un cementificio all'interno di una valle montana, in una Provincia totalmente montana e che quindi nelle sue montagne vede la sua ricchezza, non è stato mai facile, né prima dell'utilizzo del CDR-Q né oggi,

deve rispettare quelle caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche europee, leggi norme tecniche europee, leggi e regolamenti che definiscono puntualmente le condizioni e i requisiti delle operazioni di trattamento di specifiche tipologie di prodotto che solo alla fine può definirsi CSS. Sempre riportando l'esperienza personale, nella nostra azienda che produce CDR-Q c'è un'attenzione massima a questi livelli di produzione puntualmente monitorata. La produzione e l'utilizzo del CSS si inseriscono quindi nelle diverse opzioni sul processo dei rifiuti. Dai dati risulta migliorativo naturalmente rispetto alla discarica o al ricorso *tout court* all'inceneritore; non dissuade le politiche in favore della raccolta differenziata perché si tratta di lavorare un prodotto diverso rispetto a vetro, plastica, carta, umido, tutto quant'altro si può recuperare diversamente. L'utilizzo del CSS come combustibile alternativo nei cementifici è definito a livello europeo come *best available technique* (BAT), perché favorisce la riduzione di emissioni di gas serra, nonché di CO2 prodotte dalle discariche. A livello europeo - è stato ricordato prima dagli interventi - è ampiamente utilizzato: si arriva al 98 per cento in Olanda e al 61 per cento in Germania. Però, quello che non possiamo fare è convincerci solamente dell'eventuale bontà di questa pratica; riteniamo invece importante non sottovalutare oggi né mai le preoccupazioni che esprimono le comunità locali prossime agli impianti che utilizzano il CSS come combustibile nei cementifici e anche tutta la cittadinanza, soprattutto per quanto riguarda il rischio di aumento delle emissioni inquinanti,

Oggi - ho in me questa speranza e questo ottimismo - possediamo la tecnologia necessaria e le intelligenze per poterla migliorare, ovvero è ora che la ricerca e lo sviluppo tecnologico vengano impegnati per raggiungere l'obiettivo della massima sicurezza per la salute dei cittadini e per la salvaguardia dell'ambiente. Questo resta per noi il principio guida. L'articolato del nostro provvedimento è molto dettagliato, per cui ricordo solo tre punti fondamentali. la tutela della salute dei cittadini, la salvaguardia ambientale, di acqua, aria e suolo, attraverso tutti gli strumenti che abbiamo elencato, di monitoraggio puntuale sulle emissioni, di trasparenza dei dati e di confronto con la cittadinanza, di coinvolgimento degli enti locali e delle Regioni, di preciso adeguamento alle normative e agli *standard* europei. secondo punto è la revoca, da subito, di ogni atto che vada nella direzione di convertire i cementifici in inceneritori. Vogliamo evitare che vengano avviate attività imprenditoriali su questa filiera

che ha il compito di monitorare il processo della produzione del CSS e del suo utilizzo, sia attraverso strumenti volti a creare un moderno ed efficace sistema di controlli ambientali, più generalizzati e volti all'insieme ambiente, utili a garantire i livelli di sicurezza e a dare risposte sia ai cittadini che agli operatori del mercato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io voterò contro la mozione della maggioranza, non tanto perché intenda entrare nella diatriba sulla salubrità Grazie

Noi veniamo da una Regione nella quale, nella diatriba tra ciò che è ottimo e ciò che è buono, abbiamo creato vent'anni di paralisi assoluta.

Abbiamo 8-9 milioni di balle di tal quale che vengono incenerite nell'unico impianto che è stato costruito, ossia quello di Acerra, prospiciente ai Comuni di Maddaloni e di San Felice a Cancello (provincia di Caserta),

portasse surrettiziamente ad individuare i cementifici come il luogo per bruciare i rifiuti, avremmo risolto a scapito delle popolazioni della provincia di Caserta il problema della localizzazione

non di una generica possibilità di utilizzare la termocombustione nei cementifici, ma anche a guardare delle situazioni che sembrano localistiche, ma riguardano centinaia di migliaia di abitanti, che non solo sono stati penalizzati dalla installazione dell'unico termovalorizzatore, ma vedrebbero triplicati in quella zona, attraverso l'uso dei cementifici,

Qui non si tratta di migliorare la combustione del prodotto BTZ usato nei cementifici, come qualcuno vuol far passare.

In Campania abbiamo già 93 discariche piene di rifiuti tossici. Abbiamo migliaia di siti pieni di rifiuti tossici. Vuoi vedere che proprio nei cementifici di botto si brucia bene? Ma chi volete prendere per il culo?

chiamandoli signori dalla competenza non qualificata siano assolutamente inaccettabili. Non dico altro del turpiloquio, che credo non possa essere

qualsiasi senatore ha la possibilità di esprimere la propria opinione e il proprio voto in maniera insindacabile. Risponderà poi di ciò che

Mi riferisco a quei rifiuti, come ad esempio le morchie dei serbatoi e i fanghi, che diversamente non potrebbero essere smaltiti, mentre se portati a temperature alte, oltre gli 800 gradi,

avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Signor Presidente, possiamo aspettare qualche secondo, in modo da permettere ai colleghi di uscire? PRESIDENTE. Ho invitato i colleghi ad uscire con il rumore dei passi, non con il rumore della conversazione. semplicemente per portare all'attenzione dell'Aula una situazione un po' paradossale che si è venuta a creare in un piccolo comune di 11.000 abitanti in provincia di Pavia, Gambolò. Gambolò è un comune in Lomellina in cui vivono tantissime persone anziane. Durante il periodo estivo si sono trovate affisso all'entrata dell'ufficio postale un cartello con scritto: «Ufficio postale chiuso dal 5 settembre al 9 novembre per lavori».

questo paese in provincia di Pavia e diranno loro: signori, purtroppo l'ufficio postale è chiuso. Auspichiamo che questa cosa non avvenga, perché abbiamo visto che a Gambolò ci sono numerose persone anziane e l'ufficio postale più vicino si trova a parecchi chilometri di distanza.

che pagano le tasse, magari anziani che hanno lavorato una vita e che in questo momento si vedono togliere anche questo servizio, siano abbastanza indegni.

alla Camera dei deputati ad una collega era stata rifiutata la pillola del giorno dopo, in disapplicazione della legge n.

necessità, ben lieto di dare la mia prestazione in un momento così importante, perché se si parla di violenze noi interveniamo immediatamente.

Signor Presidente, ieri alla Suprema corte sono state consegnate oltre un centinaio di pagine con le motivazioni della sentenza sui fatti accaduti nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova. Le parole dei giudici lasciano di pietra, ascoltatele: «L'assoluta gravità sta nel fatto che le violenze si sono scatenate contro persone all'evidenza inermi, altre già in atteggiamento sottomissione con le mani alzate, altre dormienti» che hanno «subito una violenza ingiustificata, vendicativa e diretta all'umiliazione e alla sofferenza fisica e mentale delle vittime». Un «puro esercizio di violenza». Era stato ben compreso dai dirigenti durante le riunioni preparatorie dell'irruzione, tenutesi in questura, che l'immagine della polizia doveva essere "riscattata". Ecco, questo è stato un modo per riscattarsi. È sconvolgente. All'indomani della definitiva chiusura delle vicende giudiziarie che perdurano da dodici

incolumi anche Fini e De Gennaro, così come i dirigenti e gli agenti delle forze dell'ordine che non erano identificabili. Senza contare le 33 prescrizioni. Tra coloro che hanno pagato e sono stati condannati, Mortola, ex capo della Digos, oggi interdetto dai pubblici uffici, è riuscito nel frattempo ad essere al centro di altri episodi di violenza mentre era trasferito a capo della Polfer.

una legge sull'introduzione dei numeri identificativi sui caschi. Ma non basta! Il Governo e il Parlamento devono avviare una riforma profonda di tutto il comparto della sicurezza; introdurre criteri efficaci e meritocratici per la selezione del personale, per gli agenti e soprattutto per i dirigenti; implementare i servizi investigativi invece che militarizzare le piazze e il territorio.

parlare, signor Presidente.